Comunico che in data 14 novembre 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*: «Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti,

«farò tesoro degli indirizzi della sentenza» e poi «le opposizioni taceranno e mi auguro taceranno per sempre». del ministro Calderoli, pronunciate qualche giorno fa, dopo la decisione della Corte costituzionale di di riscrivere di fatto il disegno di legge sull'autonomia che ha portato via, colleghe e colleghi, 73 sedute della Commissione affari costituzionali - spiace che non sia in Aula il presidente Balboni

gli evidenti profili di incostituzionalità di una serie di parti di quell'impianto. Signora Presidente, non pago, il Ministro, che alcuni minuti fa a Montecitorio ha espresso parere contrario alla proposta di mozione unitaria delle opposizioni,

al presidente Malan, al presidente Romeo, al presidente Gasparri: in politica esiste un alfabeto istituzionale e poi ce n'è anche uno civile.

chiari e netti (sette per l'esattezza), mi auguro ci possa essere un momento di confronto molto serio qui in Aula; è compito di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, dire: dire: riapriamo il confronto e facciamo sì che le norme che vengono fuori - e che incidono così sulla carne viva del Paese - siano coerenti e confacenti alla Carta costituzionale. Presidente, le parole del ministro Calderoli hanno dimostrato di disprezzare sia l'alfabeto istituzionale che quello civile,

rispetto per le tesi di chi non la pensa come la maggioranza, necessità di rispettare il parere dell'opposizione; alimentare questa profonda cultura dell'insofferenza verso le regole ci preoccupa sempre di più. Pertanto, signora Presidente, noi chiediamo, attraverso di lei, al Presidente del Senato che la Presidente del Consiglio venga a riferire sulle parole del ministro Calderoli, perché vogliamo capire se quelle parole rispecchiano le parole e il punto di vista di tutta la maggioranza.

le indicazioni e le prescrizioni della Corte costituzionale, perché incideranno inevitabilmente sui lavori del Senato. Per quanto riguarda Montecitorio,

espresso più volte in Commissione affari costituzionali e in Aula - c'è sempre stato il rispetto per la forma dello Stato e per le funzioni previste dalla Costituzione che, come abbiamo ribadito più volte, poggia poggia sempre su tre principi: l'unità della Repubblica, la solidarietà, l'uguaglianza dei cittadini e le garanzie dei loro diritti. Tutti temi che sono stati violati dallo "spacca-Italia" di Calderoni. *(Applausi)*. Non vi siete fermati, perché avete deciso che i muscoli, cioè i numeri, fossero preminenti rispetto alla politica, che fossero l'unica cosa che vi interessava in quel momento rispetto al ragionamento politico. La condizione nella quale ci troviamo è questa. ve lo diciamo per l'ennesima volta. Le opposizioni sono qui che vi aspettano per riaprire il dibattito e per far sì che si torni indietro su quell'impianto, che era sbagliato. Noi continuiamo a sottolineare e a dirvi che è sbagliato. Fermatevi! Tornate qui. Cancelliamo gran parte di quella norma e proviamo a riscrivere quell'impianto, seguendo rigorosamente un'indicazione data più volte dal presidente Mattarella. L'autonomia rafforza l'unità nazionale quando attua il principio di sussidiarietà. Presidente Romeo, ciò significa attuare tutto il Titolo V, in particolar modo dall'articolo 114 al 120; non un comma, non l'articolo 116 e non l'autonomia del portafogli.

C'è un passaggio, nel dispositivo della Corte, particolarmente rilevante, ovvero quel passaggio in cui la Corte ribadisce la centralità del Parlamento nelle scelte relative all'attuazione dell'autonomia differenziata. Quest'Aula, assieme all'altro ramo del Parlamento, ha un ruolo centrale e costante nell'attuazione del Titolo V e in particolare dell'autonomia. chiediamo al Presidente del Consiglio un'informativa urgente in quest'Aula rispetto alle parole del ministro Calderoli e anche rispetto a come Governo e maggioranza intendono procedere per le modifiche di quel disegno di legge; anche a quest'Aula di ragionare, dopo quell'informativa, con delle modifiche che nascano in Parlamento, con un'iniziativa parlamentare, e non semplicemente nell'attesa di come il Governo si vorrà muovere.

del Governo. Quindi, è giusto chiedere la presenza del Presidente del Consiglio in Aula su questo tema; ma è giusto anche chiedere lo sforzo di questo ramo del Parlamento affinché si faccia parte diligente e di promozione legislativa: come sempre dovrebbe essere, ma come in questo caso è assolutamente legittimo aspettarsi.

dei presidenti Boccia e Patuanelli, sullo stesso argomento, ma vorrei iniziare il mio intervento, nella certezza di esprimere un sentimento condiviso da tutta per inviare un messaggio di vicinanza e di solidarietà a cinque militari del contingente italiano di UNIFIL

la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, proprio perché non è possibile passare sotto silenzio un duplice aspetto. Il primo è l'elemento di natura rigorosamente formale, cui si è fatto riferimento in precedenza, ossia una pronuncia della Corte costituzionale che ha stroncato, defalcato e profondamente modificato l'intero impianto di una normativa che era stata varata da questo Parlamento. Dal punto di vista strettamente procedurale, è indispensabile comprendere, anche alla luce delle dichiarazioni che il Governo ha reso nell'immediatezza del commento della sentenza, come si intenda procedere.

che noi continueremo a parlare e a dire la nostra opinione e che non ci facciamo tappare la bocca da nessuno e tantomeno dal Governo su questo, come su altri elementi. Bisognerebbe ritornare in un quadro di rispetto e di senso delle istituzioni, perché avere un Ministro della Repubblica che intima all'opposizione di tacere all'indomani di una pronuncia della Corte costituzionale è un elemento ai limiti dell'eversivo. Occorre ripristinare in quest'Assemblea, come nel Paese, l'elementare condizione di rispetto, che presuppone il fatto che in questo Paese, che è ancora una Repubblica parlamentare, con buona pace di tanta retorica, nessuno del Governo può permettersi di dire all'opposizione che deve tacere. Detto questo, siccome noi non ci spaventiamo e non ci faremo spaventare (anzi, incalzeremo nel merito il Governo su tutti questi elementi), non possiamo non far rilevare, dal punto di vista politico, la curiosità di un commento o, meglio, di una lettura arrivata dalla maggioranza. Signori della destra, sembra che questa legge sia figlia di nessuno.

un richiamo all'aritmetica, come se quei sette punti cassati non fossero il cuore della normativa, che tutta questa cosa si può fare in fretta. Fratelli d'Italia, sotto sotto, ha tirato un grandissimo sospiro di sollievo e la persona più contenta di quel pronunciamento oggi sta a Palazzo Chigi (anzi, per la verità, in questo momento sta in Brasile, ad attaccare i giornalisti italiani che hanno l'ardire di fare delle domande). *(Applausi)*. Pensate un po' a quale livello siamo arrivati. arrivati. La *Premier* sicuramente in cuor suo ha esultato per questa pronuncia e Forza Italia, che tiene un po' tutte le parti in commedia, è venuta a dire: meno male che c'è la Corte costituzionale, perché noi avevamo detto che bisognava fermarsi. Poi, però, l'avete votata. Quindi, c'è una sorta di slittamento in tutta questa vicenda che, dal punto di vista procedurale e politico, impone che il Governo riferisca in Aula.

Abbiamo passato diversi mesi in Parlamento (prima al Senato e poi alla Camera) a dire una serie di cose e a presentare diversi emendamenti nel merito. Moltissimi di quegli emendamenti evidenziavano esattamente i punti di criticità che sono poi stati affrontati giustamente dalla Corte. Ci troviamo di fronte a una sorta di stravolgimento della realtà.

vi abbiamo detto che non si poteva affrontare il tema dei LEP, così come è stato fatto nel corso dei mesi passati. Tutti avvertimenti, questi, che da parte delle forze di opposizione sono stati dati per molti mesi. a tutte queste sollecitazioni - lo voglio ricordare - nelle Commissioni competenti sia al Senato che alla Camera non sono mai state date delle risposte. Siamo davvero dinanzi a uno stravolgimento della realtà. Penso non solo che il Governo dovrebbe venire qui a riferire anche su come intende andare avanti (perché davvero non si può fare finta di niente rispetto a quello che è successo), ma penso che gli autori di questo scempio dovrebbero fare un passo indietro; lo dovrebbero al Paese, lo dovrebbero alla coesione territoriale di questo Paese e lo dovrebbero alla Costituzione italiana. Naturalmente non lo faranno, però arrivare addirittura a dire all'opposizione che non può parlare, mi sembra davvero il mondo alla rovescia. Signor Presidente, da parte nostra vogliamo assolutamente tranquillizzare le minoranze e le opposizioni, perché il confronto resta sempre aperto, così come c'è stato durante la fase di discussione della legge, della legge, che tra l'altro è rimasta in Senato, se non sbaglio, quasi un anno: era arrivata a marzo 2023 ed è stata approvata dal Senato nel gennaio 2024, con numerosi emendamenti approvati sia su proposta dell'opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. Quindi c'è stato un confronto.

vengono fatti rilievi su sette di essi, dire che la legge è stata completamente svuotata di significato, o meno,

l'autonomia si può fare: avrebbero potuto dichiarare l'incostituzionalità della legge dando sostanzialmente soddisfazione e vittoria alle Regioni che hanno fatto ricorso. In realtà l'autonomia non si ferma e la Corte dice che va avanti, ma su binari che sono differenti. Quindi vuol dire che

ci adeguiamo e ci conformiamo ai rilievi fatti dalla Corte con una discussione di carattere parlamentare, quindi con una leggina che andrà a correggere questi rilievi, poi sarà difficile sostenere che l'autonomia divide, rompe il Paese, spacca o fa tante altre cose. Voi dovete guardare un po' più avanti. Non fermatevi solo al momento politico attuale, su cui ragionevolmente fate le vostre strumentalizzazioni

a meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. Questi, di fatto, sono gli obiettivi che la Lega da sempre si propone di realizzare. Quindi, abbiamo avuto una conferma da parte della Corte del fatto che l'autonomia è funzionale e deve essere funzionale a questi obiettivi.

erano già degli obiettivi su cui già stavamo lavorando. Non si stava lavorando al trasferimento di intere materie, ma il ministro Calderoli, con le Regioni che ne hanno fatto richiesta, stava proprio lavorando per fare in modo che ci fosse un trasferimento di funzioni all'interno delle stesse materie. Questa è una conferma del lavoro che sostanzialmente il ministro Calderoli stava già facendo. Così come non penso che sia un grossissimo problema, di fatto,

avrebbe spaccato l'Italia, quello sicuramente sì. Chiudiamo con una nota lieta all'interno della stessa maggioranza: noi ringraziamo la Corte di questi rilievi eventuali, che hanno indicato dei binari

che per ora siamo in presenza soltanto di un comunicato stampa della Consulta. Tutti i costituzionalisti hanno sottolineato che, prima di decidere come procedere, è ovviamente necessario conoscere nel dettaglio le motivazioni della sentenza: quindi è necessario attendere la loro pubblicazione, a meno che il presidente Boccia e gli altri colleghi dell'opposizione non abbiano avuto modo di leggere delle anticipazioni, che però purtroppo non sono a nostra disposizione. Cosa si evince da questo comunicato stampa? Intanto una cosa fondamentale: la legge non è illegittima. La Corte ha dichiarato costituzionalmente legittima la legge, contrariamente a quanto chiedevano i ricorrenti che, in prima istanza, ne domandavano la dichiarazione di illegittimità

Ebbene, leggendo il comunicato, non sembra che queste sette norme che la Consulta ha dichiarato illegittime sconvolgano l'impianto generale della legge. Ricordo che i ricorrenti avevano sollevato qualcosa come circa 60 eccezioni di incostituzionalità. Ebbene, cari colleghi, su queste 60 eccezioni di incostituzionalità, la Corte ne ha accolte 7, ma ne ha respinte evidentemente almeno altre 53 e non sono tutte norme così fondamentali. Ne cito una soltanto: la Corte ha detto che non soltanto con norma primaria devono essere definiti i LEP, ma anche gli aggiornamenti dei LEP devono essere definiti con norma primaria, mentre come sappiamo noi nella legge abbiamo scritto che soltanto gli aggiornamenti devono essere fatti con DPCM. Non è che ci fossimo inventati questa soluzione; questa era stata presa, ad esempio, da quanto è avvenuto con la definizione dei LEA in materia di sanità. Come avviene la definizione dei LEA in materia di sanità, cari colleghi? Avviene Quindi, fermo restando l'accoglimento di queste eccezioni, che sono immediatamente applicative (perché, come sappiamo, quando la Corte dichiara incostituzionale una norma, quella norma è come se non fosse mai entrata nell'ordinamento giuridico), qual è la parte che sembra più rilevante di questo comunicato stampa e della sentenza che siamo tutti curiosi di leggere? È la parte in cui la Corte non dichiara l'illegittimità di altre norme, ma dice che possono essere ritenute legittime a condizione che siano interpretate in senso costituzionalmente orientato. È chiaro a tutti che per capire esattamente la portata di questa terza parte della sentenza sia assolutamente necessario poterla leggere. Vi garantisco che quando avremo a disposizione la legge, come maggioranza, faremo in modo di seguire - perché questo è dovere del Parlamento - le indicazioni della Corte costituzionale. Sinceramente non capisco lo scandalo, non capisco nemmeno l'esultanza dell'opposizione: il dato di fatto è che la Consulta ha dichiarato legittima la legge la legge e ha detto che essa è assolutamente necessaria perché garantisce maggiore efficienza e soprattutto l'applicazione del principio di sussidiarietà, che voi avete inserito nel Titolo V della Costituzione per lasciarlo inattuato per ventidue

mi consenta un richiamo al privilegio dell'età. Ventitré anni fa in quest'Aula si tenne una battaglia parlamentare memorabile, durata tre giorni, per approvare la riforma del Titolo V. Il privilegio dell'età fa sì che, non avendo perduto ancora completamente la memoria, ricordi bene quei giorni ricordo bene anche la battaglia sull'articolo 116, comma 3. Ora, pazienza per quelli che, come il senatore Borghi e il suo Gruppo, non erano ancora nati. Pazienza ugualmente per il senatore Patuanelli e il suo Gruppo che non erano ancora nati: ma il senatore Boccia, se non ricordo male, aveva già fatto la prima comunione,

partiti tradizionalmente federalisti e regionalisti trovarono il supporto insperato del partito del senatore Boccia.

coloro, che sono i responsabili primi di quella riforma costituzionale, oggi stiano cercando, e abbiano cercato durante l'approvazione di questa misura, di coprire lo scempio costituzionale che fu fatto allora Ci potremmo parlare con un po' più di pacatezza e vedere quali sono questi punti; comprendere se veramente essi sono fondamentali ed essenziali; essenziali; se contribuiscono al meglio all'efficienza del sistema amministrativo e legislativo italiano; se spaccano o meno l'Italia - come è stato detto - oppure dobbiamo continuare ancora a fare propaganda come quella che abbiamo e stiamo facendo oggi? La sto facendo anche io: mi

luminare della questione, che molto appassionatamente indicava i punti deboli della riforma, che però non furono ascoltati. Se non ricordo male, soltanto tre o quattro voti di maggioranza fecero sì che questa riforma storica passasse. Oggi la vogliamo coprire con una leggina ordinaria: ci vergogniamo dello scempio e la nascondiamo? Non mi pare serio, perché il tema è di grande momento storico storico e costituzionale. Qui si sta toccando un tema che fu lungamente e approfonditamente dibattuto nell'Assemblea costituente:

intervenuta e vediamo che cosa si può fare, lasciando la campagna elettorale su questo punto ad un altro momento. Grazie per l'appello al privilegio.

il presente disegno di legge di iniziativa governativa deriva dallo stralcio da parte della Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato, dell'articolo 23 del disegno di legge Atto Senato 1184, 1184, deliberato per estraneità del medesimo articolo 23 all'oggetto del suddetto disegno di legge. Il disegno di legge n. 1184-*bis* autorizza il Ministero della salute ad assunzioni ad assunzioni con contratto a tempo determinato aventi scadenza non successiva al 31 dicembre 2025 di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero. La finalità delle nuove assunzioni è costituita dal potenziamento delle attività di vigilanza, controllo igienico e sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti e al conseguimento di un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie, derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che partecipano al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. Il disegno di legge reca anche le autorizzazioni di spesa relative alle assunzioni in oggetto e la corrispondente copertura finanziaria. Le assunzioni autorizzate dal disegno di legge concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni in oggetto devono riguardare soggetti che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo, sino al 31 dicembre 2023 e per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

superamento di apposite procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, su base regionale, che prevedevano, al termine del periodo di prova, il superamento di un ulteriore esame teorico-pratico, quale condizione per la conferma dell'assunzione. Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, autorizzò il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione. Le assunzioni potevano essere effettuate utilizzando graduatorie - sia del medesimo Ministero sia approvate da altre amministrazioni - per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale; al termine del periodo di prova, a cui erano soggetti anche coloro che lo avessero già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione era subordinata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. La finalità delle assunzioni era costituita dal potenziamento - anche in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - delle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti. Le autorizzazioni di spesa poste dal presente disegno di legge sono distinte con riferimento agli emolumenti per il personale (ad esclusione delle voci qui successive), all'erogazione dei buoni pasto e ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario. In sede redigente, gli importi relativi all'anno 2024 sono stati ridotti, in considerazione del ridotto periodo di tempo che può intercorrere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2024. Alla copertura corrispondente alle suddette autorizzazioni di spesa si provvede mediante riduzione - negli importi complessivi annui ivi indicati - dell'autorizzazione di spesa relativa alle "transazioni da stipulare con soggetti talassemici o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti".

Presidente, colleghe, colleghi, anche se il provvedimento sembra sembra limitato, in realtà riguarda un evento storico, perché davvero il Giubileo della Chiesa cattolica ogni volta cambia i fogli della storia, magari non direttamente, magari in maniera indiretta, ma spesso - per fortuna - diretta, aumentando i diritti - scusate il giro di parole - la rappresentatività e la consistenza dell'anima sulla concretezza della quotidianità. Quest'anno, con molta lungimiranza, ma anche con un po' di rischio, il Santo Padre Francesco aprirà due porte, una nella sede logica logica e storica, un'altra nel carcere romano, per rappresentare che il Giubileo riguarda tutti, anche le cosiddette anime perse, che non lo sono mai, perché c'è sempre speranza nella redenzione, nel tornare indietro, nel rappresentare l'orrore dei propri delitti con la voglia di riscatto. In questa realtà, dove purtroppo troppi cittadini si arrabbiano per i lavori che hanno portato al Giubileo, per i disservizi momentanei, per le difficoltà di

poter garantire prevenzione, diagnosi precoce, cura ed eventuale riabilitazione, traguardando la realtà di salute, di sofferenza o addirittura di malattia, attraverso chi arriva dai porti o dagli aeroporti, credo sia un viatico di enorme significatività. È un Giubileo che si occupa, con molta attenzione - direi santa - delle anime, ma che non trascura il corpo, non trascura il momento di prevenire, curare, riabilitare.

non voglio avere l'arroganza di dire che solo io ho questo dono rispetto a tante persone che non credono, anche se credo poco che la gente non creda, magari nel chiuso della propria anima. Credo che poche volte abbiamo fatto una proposta lungimirante, seria, che è anche un modello di intervento politico, tecnico, scientifico, ma anche emozionale rispetto al raddoppio della popolazione in Italia per un periodo lungo - un anno, poi ciascuno starà un giorno o tutto l'anno

una mossa, o comunque una scelta - mettiamola così- che in qualche modo determina la lesione del diritto di qualche categoria sociale. Dico questo apertamente, molto chiaramente e anche con un grado di indignazione molto elevato, signora Presidente. Ovviamente noi sappiamo che c'è il Giubileo: ce ne siamo già occupati in Parlamento più di una volta, abbiamo votato una serie di provvedimenti. Quindi, un evento e di una circostanza noti e prevedibili, di cui si discute già da tempo. Ed ogni istituzione è chiamata a fare la sua parte in termini di spesa, in termini di programmazione dei lavori e in termini di calendarizzazione degli stessi, in termini di obiettivi da raggiungere, in termini di controlli sanitari nei porti e negli aeroporti. Questo perché il numero dei pellegrini attesi a Roma per l'anno giubilare 2025 è altissimo e sicuramente ci sarà necessità di intensificare i controlli e di garantire la presenza di personale medico. Ma qui, evidentemente e come sempre, siamo davanti all'approssimazione di questo Governo, che intanto si muove sempre sul fil di lana ed arriva a portare in Aula questo provvedimento oltre la metà del mese di novembre del 2024, con le assunzioni da da farsi entro il 2025 per l'anno giubilare: quindi, siamo sempre alla prossimità della scadenza degli interventi da adottare. Poi, come sempre, non ci sono una visione, una programmazione, ma vi è sempre una misura urgente, una necessità di intervenire *in limine litis* per adottare un provvedimento che, in questo caso, prevede l'assunzione di tre dirigenti sanitari medici e di quindici funzionari con profilo tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Quindi, stiamo parlando di un numero ridotto, di una consistenza numerica non elevatissima. a fronte della evidente non grandezza dei numeri delle assunzioni a tempo determinato - per la durata di un anno, da scegliersi tra personale medico che abbia svolto già servizio presso il Ministero per almeno tre anni alla data del 31 dicembre 2023 - è chiaro che stiamo individuando una categoria di lavoratori già predefinita. Non ci stiamo rivolgendo a tutti i dirigenti sanitari che esistono in Italia e a tutti i funzionari con profilo tecnico. Ci stiamo rivolgendo a quelli che già hanno svolto servizio presso il Ministero. Ma se dovevamo fare questo intervento, se dovevamo rimpolpare le fila dei dirigenti sanitari e dei funzionari tecnici, credo che, prima di fare un disegno di legge - prevedendo l'assunzione di diciotto unità, si poteva procedere con interpello; si poteva procedere con la mobilità interna; si potevano, cioè, attivare tutte quelle misure che già esistono nella pubblica amministrazione. In virtù di queste procedure, quando ci sono straordinarie esigenze e necessità, si può attingere dal personale che già opera dentro l'amministrazione, che già è assunto, che già è alle dipendenze. Normalmente, ci viene insegnato che, solo quando l'interpello non si conclude con esito favorevole e non c'è la possibilità di attingere al personale già esistente, si ricorre alla via straordinaria di un'assunzione a tempo determinato. Pronuncio il termine "determinato" scandendolo chiaramente, perché già l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea per il ricorso al lavoro a tempo determinato in assenza di specifiche prescrizioni e in assenza di giustificazioni che legittimino questa forma di lavoro. Ricordiamo sempre, perché l'Europa ce lo ha rammentato e ci ha sanzionato per questo, che il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato e che solo per straordinarie esigenze, che devono essere motivate, si può fare ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato. Voi vedete straordinarie esigenze? No: nella misura in cui sapevamo già da un po' che c'era il Giubileo e potevamo prevedere, già prima, di assumere il personale necessario. Straordinarie esigenze per reperire questo personale? No: potevamo prevedere di reperirlo in altro modo e poi, forse, solo dopo aver documentato l'impossibilità di assumerlo in questo modo, accedere a una forma straordinaria di assunzione a tempo determinato delle diciotto unità di personale; che, peraltro, vengono scelte non nella selezione universale dei lavoratori del comparto della sanità, ma soltanto fra quelli che hanno già prestato servizio presso il Ministero. Quindi, creiamo una categoria già di elezione presso la quale facciamo tali assunzioni. rilievi, signor Presidente, che potrebbero anche essere superati, semplicemente accettando che purtroppo i governanti sono approssimativi e miopi, per cui va posto rimedio in qualche modo alla loro disattenzione costante e cronica verso i provvedimenti da adottare, vi

per l'anno 2025, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La maggior parte di noi ha sentito questi numeri e ha pensato: li hai letti, brava. Ma questi numeri, per chi appartiene alle categorie tutelate da questa legge, sono gravi.

affetti da emoglobinopatia, emofilici, emotrasfusi, danneggiati da trasfusioni di sangue infetto o da emoderivati, o soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

che hanno un giudizio pendente. Noi togliamo quindi risorse a chi ha un danno certo e ha chiesto di ottenere un indennizzo. Nel fare la relazione e nel dare il parere

indennizzare i soggetti che hanno avanzato una domanda di risarcimento del danno nei confronti del Ministero della salute per trasfusioni occasionali o per danni permanenti alla loro integrità fisica Come anticipato, non vorrei essere mai nei panni di quel soggetto che, dopo aver intentato un giudizio e dopo tutte le lungaggini del procedimento in Italia, magari dopo dieci anni di attesa, ottiene finalmente una sentenza di condanna con liquidazione di un indennizzo e, quando promuove l'azione per ottenere il risarcimento del danno (ossia, la liquidazione, il ristoro, né più né meno di quello che gli serve soltanto per ristorare il danno economico), si sente rispondere dal Ministero che, in quel momento, quelle somme non sono disponibili perché il fondo è stato estinto, o comunque ridotto per effetto di provvedimenti come quello

a rimpinguare e restituire le risorse necessarie sul fondo nel primo intervento di bilancio possibile. Ciò non si legge in questo provvedimento e non è previsto nella legge di bilancio.

l'assunzione di 3 dirigenti e 15 funzionari a tempo determinato, per l'anno 2025,

sono migliaia le persone che sono in contenzioso su questo terreno. Non abbiamo idea di quanto possa costare e rispondere adeguatamente alla richiesta delle persone coinvolte, intanto però si attinge. E credo che non sia solo questo il fondo in cui c'è disponibilità. Questa è la sottolineatura che noi vogliamo fare. In sostanza, siamo di fronte a una situazione di questo genere e spostare le risorse ci pare del tutto sbagliato e ci lascia un po' l'amaro

il disegno di legge in esame rappresenta una risposta a un problema di carenza temporanea di personale sanitario e amministrativo, che viene ora risolto. Nella legge di bilancio è previsto l'aumento graduale delle risorse per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale porterà la dotazione dai 134 miliardi del 2024 ai 144 miliardi del 2030. 2030. Tali stanziamenti sono cresciuti anche in rapporto al PIL rispetto all'anno pre-Covid e - come abbiamo tutti avuto modo di vedere - continuano a crescere. Parte di queste risorse serviranno a razionalizzare la sanità pubblica, dove pure persistono delle sacche di inefficienza. Ricordiamo inoltre che in questo momento è in azione il PNRR, che prevede una riforma complessiva dell'assistenza medica territoriale; pensiamo all'introduzione della telemedicina e all'adozione dei fascicoli sanitari elettronici. È vero: rimane il grande tema della carenza di personale medico e infermieristico, cui però si sta mettendo mano con altri provvedimenti; tra questi, la riforma delle professioni sanitarie, che determinerà un nuovo modo di approcciare le cure sanitarie. Va fatto un plauso soprattutto alla riforma degli accessi alla laurea in medicina, fortemente voluta dalla ministra Anna Maria Bernini. Nel frattempo registriamo che si supplisce alla carenza di medici e di infermieri attingendo a professionalità che provengono dall'estero;

Paesi europei, perché ovviamente le viene garantita una migliore condizione economica. Si tratta di una serie di problemi, Presidente, che va risolta in modo strutturale. Ci sono le competenze, sia al Governo che in Parlamento, per affrontare in modo completo queste tematiche.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, oggi siamo chiamati a votare il disegno di legge n. 1184-*bis*, un provvedimento in vista del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. mira a garantire la sicurezza sanitaria dei milioni di pellegrini attesi. È nostra responsabilità, come legislatori, assicurare che il Sistema sanitario nazionale possa rispondere in modo adeguato a eventi di tale portata e il disegno di legge in discussione permette di affrontare questa sfida. L'autorizzazione ad assumere nuove unità di personale provenienti da un contesto professionale già consolidato nel Ministero della salute rappresenta una scelta rispettosa delle competenze, sebbene a tempo determinato. Va da sé che la presenza a tempo determinato di dirigenti sanitari, medici e tecnici della prevenzione potrà contribuire ad innalzare i livelli di protezione della salute pubblica per un breve periodo, quando però il nostro primo obiettivo di salute pubblica sarebbe quello di garantire e aumentare in modo strutturale le piante organiche della sanità pubblica. Voglio sottolineare che, riguardo alla copertura degli oneri finanziari, il MoVimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti al Governo, che sono arrivati. È evidente però che la scelta di attingere risorse dai fondi già destinati ai risarcimenti per i soggetti danneggiati dalle trasfusioni abbia suscitato delle preoccupazioni. Pertanto è stata nostra premura assicurarci che i diritti di queste persone non siano compromessi da scelte che, sebbene fondate su situazioni di necessità, possono sembrare poco trasparenti. Per noi la salute dei cittadini deve rimanere la priorità. A causa di queste perplessità in merito alla copertura economica e alla logica dietro ad alcune scelte - riteniamo

Ne ha facoltà. MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, colleghi e colleghe, il Giubileo del 2025 rappresenta un'occasione straordinaria per la nostra Nazione. È quindi necessario predisporre tutti gli opportuni interventi per prepararsi ad accogliere al meglio i circa 30 30 milioni di pellegrini che giungeranno nella capitale e nelle altre Province del Lazio, affinché questo evento così importante possa essere vissuto nel massimo della sicurezza. Il Governo e la Regione Lazio, in modo sinergico, stanno lavorando moltissimo per questo. Proprio sulla scorta di tale necessità è stato presentato dal Governo il disegno di legge n. 1184-*bis*, il quale deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato dell'articolo 23 il quale autorizza il Ministero della salute ad assunzioni con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero. La finalità delle nuove assunzioni è costituita dal potenziamento dell'attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, ed al conseguimento di un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Il disegno di legge reca anche le autorizzazioni di spesa relative alle assunzioni in oggetto e la corrispondente copertura finanziaria. autorizzate dal disegno di legge n. 1184-*bis* concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni in oggetto devono riguardare i soggetti che abbiano già presentato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023 e per almeno quindici mesi con contratti di lavoro a tempo determinato. 17 marzo 2020, n. 18, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenente

Le autorizzazioni di spesa, invece, poste al presente disegno di legge, sono distinte con riferimento agli emolumenti per il personale, all'erogazione dei buoni pasto e ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario. In sede redigente, gli importi relativi all'anno 2024 sono stati ridotti in considerazione del ridotto periodo di tempo che può intercorrere tra l'entrata in In linea con le finalità del presente disegno di legge si pongono le iniziative a livello regionale in ordine all'assunzione di personale, all'acquisto di nuovi macchinari, alla revisione della programmazione dei pronto soccorso al fine di renderli più efficienti, più accoglienti e potenziati, all'implementazione delle ambulanze, auto mediche e defibrillatori. È importante quindi la macchina messa in campo per l'assistenza sanitaria ai milioni di pellegrini che arriveranno nella Capitale per il Giubileo che si aprirà il 24 dicembre. 34 gli interventi complessivi dati dalla Regione per potenziare il servizio sanitario regionale, per un totale di 155 milioni di euro di investimenti, di cui circa la metà, vale a dire 70 milioni, soltanto per Roma. Tale disegno di legge è dunque essenziale, poiché si pone in combinato disposto con gli interventi predisposti anche a livello regionale, per affrontare questo evento così importante per il nostro Paese. Per tali motivazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. Mi permetta, Presidente, però di sottolineare

per continuare a sbloccare servizi e trasporti a piacimento, anche durante il Giubileo. Questa è solo una furia ideologica della CGIL contro il Governo, ma ne pagheranno direttamente le conseguenze tutti i settori e l'immagine del nostro Paese. Quindi, chiedo al presidente Landini di andare a rivedere anche la sua posizione, perché il protocollo d'intesa per il Giubileo va direttamente a salvaguardare anche la sicurezza dei pellegrini.

di un disegno di legge che prevede, come è stato ricordato, l'assunzione fino al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo determinato di tre dirigenti sanitari medici e di 15 tecnici della prevenzione, con esperienza di almeno quindici mesi. Si tratta evidentemente di un provvedimento che ha un senso e che per chi, come me, ha vissuto in prima persona l'emergenza Covid; è evidente che poter avere un rafforzamento dei controlli sanitari, nel momento in cui il nostro Paese verrà raggiunto da migliaia e migliaia di pellegrini da tutto il mondo, è necessario ed importante. Peccato, però, che questo provvedimento, apparentemente innocuo, nasconda alcuni errori e alcune mancanze politiche molto serie. anzitutto il punto che prevede per l'ennesima volta assunzioni a tempo determinato, che devono rispettare i limiti triennali previsti.

il Giubileo sia un'emergenza. Tutti sapevamo che arrivava il Giubileo e tutti sapevamo in quale anno sarebbe stato celebrato. Non si può quindi di nuovo argomentare che l'emergenza costringe il Ministero ad assunzioni a tempo determinato. Sarebbe veramente venuto il momento di superare queste modalità; tra l'altro, come è stato ricordato, si tratta di assunzioni con procedure non proprio trasparentissime. Troviamo

che si possano sottrarre i soldi o comunque impiegarli per fare altro. Quei soldi vanno messi a fare esattamente quello, magari in un capitolo di spesa di un anno successivo. Riconosciamo e ci assumiamo naturalmente anche noi, come è giusto che sia, l'esercizio della responsabilità rispetto alla necessità di accertamenti sanitari rafforzati e maggiorati per il Giubileo 2025. Tuttavia, per le modalità utilizzate e anche per il fatto che, essendo novembre, parliamo di una cosa che praticamente è dietro l'angolo, perché tutto questo parte a gennaio 2025,

Come è noto, il disegno di legge in discussione è la risultante dello stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184 che riguardava disposizioni per la semplificazione in materia di attività e servizi ai cittadini. In esso sono contenute misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del prossimo Giubileo della Chiesa cattolica, che si aprirà ufficialmente la sera del 24 dicembre con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro. Il Giubileo rappresenta certamente un evento planetario, una grande sfida, ma anche una grande opportunità per l'Italia e per Roma, con la previsione dell'arrivo di 35 milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo: un numero maggiore di quanti ne furono registrati nelle due precedenti occasioni, rispettivamente nel 2000, quando furono quasi 33 milioni, e del Giubileo straordinario del 2015, con circa 23 milioni di presenze. Ripercorrendo il significato e il valore del Giubileo, ricordo che esso trae le sue origini dalla tradizione ebraica: ogni cinquant'anni gli ebrei decretavano un anno di riposo dei campi allo scopo di far riposare il terreno e renderlo più fertile per la stagione successiva. Contemporaneamente, gli schiavi venivano liberati e le terre confiscate venivano restituite in modo che le diseguaglianze fossero appianate. Anche il nome stesso del Giubileo ha un'etimologia ebraica: la parola ebraica *jobel* indica infatti il caprone, il cui corno veniva suonato per indicare l'inizio del Giubileo. Il primo Giubileo della Chiesa cattolica fu proclamato nel 1300 da Papa Bonifacio VIII. Per la prima volta veniva concessa l'indulgenza plenaria a tutti coloro che avessero fatto visita alle basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le mura, probabilmente sulla scia della Perdonanza celestiniana nel 1294. Questo evento viene ricordato da Dante nel XVIII Canto dell'Inferno, dove, descrivendo l'enorme flusso di pellegrini, egli paragona il procedere in senso opposto delle due schiere di peccatori della prima bolgia ai pellegrini che sul Ponte Sant'Angelo, durante il Giubileo, si incrociavano gli uni diretti a San Pietro, gli altri - di ritorno - diretti a Monte Giordano. Dal 1300 sono stati indetti 29 giubilei, l'intervallo è cambiato più volte nel corso della storia secolare, ma oggi è di venticinque anni; l'ultimo Giubileo ordinario è stato quello del 2000, che segnò l'inizio del terzo millennio. Il Giubileo ha per i cattolici un profondo valore spirituale: infatti comunemente viene detto "anno Santo", non solo perché inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri, ma anche perché è destinato a promuovere la santità di vita. Papa Francesco, quando ha annunciato, con la bolla di indizione, il Giubileo ordinario della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ha voluto dare un segnale e un messaggio di speranza, un'occasione di rinascita dopo le sofferenze che hanno segnato l'umanità negli ultimi anni, rammentando le radici di questo momento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale, che nel corso dei secoli ha rappresentato un dono di grazia per tanti fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, con le indulgenze e testimonianze vive di fede. opportunità, una grande vetrina, ma anche una prova importante per Roma, cuore dell'evento, che dovrà dimostrare di essere una città funzionale e accogliente, sostenibile e inclusiva e dove è prevista la realizzazione di opere e di iniziative di sviluppo, con un'attenzione particolare alle periferie della città. Ci sono oltre 1.000 cantieri aperti per più di 200 progetti, tra i quali la riqualificazione di Tor Vergata che, insieme al quartiere Centocelle, ospiterà alcuni degli eventi più importanti del Giubileo, la riqualificazione di Piazza San Giovanni in Laterano; altri importanti progetti sono previsti per migliorare la viabilità, come la realizzazione del sottopasso di Piazza Pia, un tunnel che dovrebbe alleggerire il traffico, consentendo la ridefinizione di un'area pedonale tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione fino a piazza San Pietro, e molto altro ancora. Ritornando al disegno di legge che ci accingiamo a votare, si prevede che il Ministero della salute sia autorizzato ad assumere - con contratto di lavoro a tempo determinato e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025 - tre dirigenti sanitari medici e 15 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Si tratta di personale che ha già maturato una significativa esperienza nel settore dei controlli e ha acquisito competenze che contribuiscono a garantire il buon funzionamento degli uffici periferici, con le prime frontiere, nel contrasto alla diffusione degli agenti patogeni. La presenza di questo personale presso gli uffici periferici è necessaria per lo svolgimento delle delicate attività di profilassi internazionale e sorveglianza sanitaria nei principali porti ed aeroporti, a tutela della salute pubblica, in considerazione dell'esigenza di assicurare tempestivamente l'erogazione dei servizi all'utenza e aumentare l'efficienza delle strutture di fronte al grande incremento dei flussi di ingresso sul territorio nazionale legato al Giubileo. Pertanto, con questa proposta normativa, si mira a potenziare la funzionalità degli uffici periferici, ad adeguare i servizi al flusso di utenza previsto per il Giubileo, consentendo al Ministero della salute di rafforzare le proprie strutture senza disperdere la professionalità acquisita dal personale già impiegato per queste funzioni. Per quanto riguarda, poi, la decurtazione dei fondi dedicati ai talassemici e agli emotrasfusi, ricordo che, a seguito del DPCM del 26 maggio 2000, le funzioni di indennizzo sono trasferite alle Regioni, tranne che per la Regione Sicilia. il Ministero ha una spesa fissa per 9.000 indennizzi per circa 90 milioni su un capitolo di 240 milioni. Mi sento quindi di rassicurare, perché la riduzione non pregiudica le finalità a cui sono destinati i fondi per gli indennizzi. In conclusione, colleghi, il contenuto del disegno di legge rappresenta un utile contributo per garantire il buon funzionamento delle strutture di sorveglianza sanitaria in vista di questo importante evento, pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Signor Presidente, la relazione sarà condivisa con la senatrice Minasi,

sono la velocità di autoveicoli e motoveicoli, la distrazione, anche legata all'utilizzo del telefono cellulare, la guida in stato di ebbrezza

alcuni degli ordini del giorno già approvati in Commissione hanno un valore d'impegno rispetto quello che sarà poi l'intervento del Governo e la successiva delega.

Importante è anche l'articolo 2, che inasprisce il quadro sanzionatorio per quanto riguarda l'abbandono di animali, stabilendo che le pene per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali si applichino anche quando questi eventi dipendano dall'abbandono di animali per strada. L'articolo 3 introduce una nuova disciplina, quella dell'alcolock, che è un dispositivo che sostanzialmente impedisce l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero per i guidatori recidivi dal punto di vista dell'utilizzo di sostanze alcoliche oltre i limiti consentiti. L'articolo 4 modifica, rendendolo più rigoroso, il sistema di penalizzazione del punteggio sulla patente, introduce la sospensione breve della stessa e inasprisce il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità all'interno del centro abitato e per l'uso dei telefoni durante la guida. Vi è poi l'articolo 5, che prevede una sorta di premialità per chi partecipa a corsi extracurricolari e di educazione stradale, organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e dalle autoscuole. Costoro avranno un credito di due punti per il rilascio delle patenti di vario genere. L'articolo 6 introduce il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza sulla circolazione dei mezzi di trasporto. L'articolo 7 interviene sulle limitazioni di guida per i neopatentati, con un aumento della potenza dei veicoli, ma al contempo, in relazione ad alcune necessità evidenziate nell'esame alla Camera, estendendo la durata del limite da uno a tre anni. Quindi, da questo punto di vista, intervenendo anche sulla limitazione e il controllo della guida dei neopatentati. L'articolo 8 introduce ulteriori obblighi relativi alle esercitazioni alla guida, in particolar modo prevedendo l'obbligo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane, anche in condizioni di guida notturna, come *conditio sine qua non* per proseguire con la certificazione da parte dell'autoscuola, e quindi la la possibilità di svolgere regolarmente le esercitazioni. L'articolo 9 abbassa i limiti di età per condurre i veicoli adibiti al trasporto di persone a favore dei titolari di carta di qualificazione del conducente. L'articolo 10 apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico. Nel caso di

il cumulo materiale delle sanzioni, quindi si tratta di una nuova disciplina sul cumulo, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove favorevole. Per quanto riguarda l'articolo 11, specifico per la città di Venezia, introduce apparecchiature di rilevamento per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua. L'articolo 12 disciplina le campagne di richiamo dei veicoli per i quali sia stata rilevata la presenza di un rischio grave. L'articolo 13 prevede una nuova disciplina dei compensi per il personale della motorizzazione civile. L'articolo 14 introduce per la prima volta una disciplina precisa sui monopattini. Si prevede, tra le altre misure, l'obbligo di esporre un contrassegno identificativo, l'obbligo del casco per tutti i conducenti, l'autorizzazione a circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 chilometri e l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Chiediamo quindi anche qui di intervenire su un tema fino ad oggi non adeguatamente normato. Si introducono, inoltre, sanzioni per chi circola con un dispositivo di micro mobilità elettrica diverso dai monopattini, con caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle che, con apposito decreto ministeriale, sono definite. L'articolo 15 reca poi una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, con la modifica di alcune definizioni legislative, dei poteri dei Comuni di regolamentare la circolazione nei centri urbani e della disciplina della precedenza e del sorpasso, nell'ottica di una maggiore tutela di chi conduce biciclette. Si prevede, inoltre, Si prevede, inoltre, l'inclusione dei conducenti di ciclomotori e di motocicli tra gli utenti vulnerabili della strada. di un divieto di circolazione dei motocicli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a favore di alcune tipologie di motocicli, a condizione che siano condotti da un soggetto di maggiore età. l'articolo 17 si modificano le norme di comportamento per quanto riguarda i conducenti in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, anche qui nell'ottica di una maggiore sicurezza stradale. L'articolo 18 reca poi misure volte a facilitare l'attraversamento pedonale delle persone che abbiano disabilità visiva. Infine, per quanto riguarda la mia parte di relazione,

Voglio sottolineare quanto in questo momento sia importante il tema della sicurezza. Anzi, direi che soprattutto oggi sta diventando un'emergenza perché non possiamo più tollerare o restare fermi davanti ai tanti giovani che perdono la vita sulla strada. Siamo convinti che questo complesso di norme, che sicuramente non potrà azzerare gli incidenti stradali, potrà consentire, con regole

misure di regolazione dei flussi veicolari volti a proteggere gli operatori stradali e prevenire situazioni di pericolo sulla carreggiata, mentre l'articolo 21 prevede che i segnali luminosi di pericolo e i segnali a messaggio variabile debbano essere debbano essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificare il momento di accensione e spegnimento e il regolare funzionamento.

L'articolo 25 dispone che possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale in tutti gli ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO. L'articolo 26 fissa un tetto massimo alla maggiorazione dovuta in caso di ritardato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal codice della strada. Tale tetto non può mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione. sanzione. L'articolo 27 circoscrive i poteri dei sindaci di limitare la circolazione nei centri abitati ai casi in cui questo risulti strettamente necessario e tenuto conto delle esigenze della mobilità. Con infrastrutture e dei trasporti saranno individuate le tipologie dei Comuni che possono avvalersi di questa facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni, nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare nelle aree oggetto di limitazione, per evitare di arrecare disagio ai cittadini. L'articolo 30 estende la possibilità di utilizzare autobus locati senza conducente da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada, al fine di ovviare alla carenza di autisti. L'articolo 35 reca delega al Governo, da esercitare entro dodici per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e circolazione. Lo stesso articolo, poi, autorizza il Governo a emanare regolamenti di delegificazione della disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli l'aggiornamento della segnaletica stradale (anche questo importantissimo). L'articolo 36 prevede che il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possa aggiornare il regolamento di attuazione del codice della strada. Infine, è presente la clausola di invarianza finanziaria. Mi auguro che questo disegno di legge possa trovare in Assemblea la stessa condivisione manifestata in Commissione. Ringrazio tutti i componenti della Commissione e il presidente Fazzone, perché credo che questa legge di riordino possa davvero rappresentare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza delle nostre strade.

la strategia di questa maggioranza e soprattutto di questo Governo, in specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verso una maggiore sicurezza e un aggiornamento del quadro normativo di riferimento del mondo che viaggia, della parte della comunità che si sposta quotidianamente con mezzi propri lungo le strade delle nostre città, lungo le nostre autostrade e lungo tutto quel grandissimo reticolo di viabilità che sin dall'antichità caratterizza la comunità nella quale viviamo.

Devo dire e lo ripeto: pochi giorni fa sono intervenuto per lodare questa maggioranza che ha avuto il mandato popolare per esprimere dei convincimenti che sono alla base del consenso che abbiamo ricevuto nelle passate elezioni politiche, e per portare avanti quel quadro di riforme, soprattutto relative alla sicurezza dei cittadini, che gli elettori ci hanno puntualmente richiesto di attuare. Oggi parliamo quindi della sicurezza stradale e, rifacendomi ancora alle parole di colui che è il mio *leader* di partito, ma è anche ministro e Vice *Premier* di questo Paese, Matteo Salvini, chi non c'è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti. Voglio partire da qui, da coloro che - ahimè - sono vittime di quei fatti che quotidianamente accadono sulle vie pubbliche e che purtroppo

avevano davanti a sé un futuro che viene distrutto dagli eventi che sono quotidianamente e reiteratamente sotto gli occhi di noi che dobbiamo leggere di queste tragedie ogni giorno sulla stampa. Partirò da uno di loro perché proprio il Vice *Premier* ha potuto parlare con la madre del defunto Stefano Sanna,

si è trovato di fronte sulla stessa corsia, ma in senso opposto (quindi contromano), un'autovettura guidata da un automobilista ubriaco che è stato trovato con un tasso alcolico ben sette volte superiore al limite di legge. nello scontro Stefano è morto e la madre Sara, coraggiosamente, ha voluto portare avanti una battaglia. Io la ringrazio perché ci siamo incontrati anche in quel di Siena, proprio con il ministro Salvini, e grazie a questa interlocuzione nasce oggi, in questo testo, l'articolo 22 per il contrasto del rischio della circolazione contromano. È una sperimentazione di cui abbiamo fortemente parlato al ministro Salvini e che trova oggi in questo provvedimento una risposta che vedrà, per la prima volta in Italia, questo tipo di tecnologie aiutare a prevenire altre stragi sulle nostre strade. strade. Non sappiamo infatti chi potrebbe trovarsi domani sulla strada, quando un disgraziato, che può tra l'altro anche beneficiare di una pena patteggiata, si potrebbe mettere nuovamente alla guida e distruggere altre vite. È con questo spirito che nasce il testo normativo che ci accingiamo a votare e a far diventare finalmente legge dello Stato. Qualcuno ha parlato di Governo della sicurezza e di un codice repressivo.

Abbiamo veramente una varietà molto articolata di norme. Il primo punto, su cui abbiamo fortemente combattuto, è quello che riguarda l'uso di droghe o di sostanze alcoliche. Per quanto riguarda l'uso delle droghe, c'è una grande semplificazione per le Forze di polizia: gli organi accertatori non dovranno più verificare la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica. Un'altra norma che abbiamo fortemente voluto è frutto di una diversa sensibilità, che nella nostra comunità trova molto riscontro: la pericolosa condotta dell'abbandono degli animali lungo le nostre strade, che spesso può causare involontariamente anche morti e feriti. Per coloro che si trovano ad abbandonare animali lungo le vie pubbliche

si arriverà a comminare delle pene molto pesanti e sicuramente social-preventive. dopo decenni di attesa e dopo troppe tragedie, figli di una distrazione e di un'imprudenza che probabilmente è anche il frutto dell'incapacità della nostra società di trovare dei momenti di formazione idonei a prevenire nei giovani quelle tentazioni adolescenziali a causa delle quali si vuole sfidare la sorte, si vuole sfidare la fortuna, si vuole essere gradassi. Questi comportamenti purtroppo mettono a serio rischio la vita

di trasformare questa società in uno Stato più sicuro, più responsabile, maggiormente parco di fronte a quei comportamenti che, guarda caso, nella maggior parte dei casi sono causa di tragedie.

del ritiro del titolo di guida. Su questa norma abbiamo molto studiato (era una mia proposta di legge nella passata legislatura) per cercare di aumentare il tempo utile, anche perché, con una sospensione di sei mesi, mesi, un lavoratore stagionale potrebbe non ingiustamente trovarsi impossibilitato a richiedere immediatamente il permesso orario. un termine, che riteniamo congruo, di quindici giorni dal momento del ritiro per richiedere un permesso orario; ci sembra una norma di buonsenso. Vado a concludere ricordando anche quelle

inciso da precedenti sanzioni. Possiamo certamente anticipare il nostro favore per questo compendio normativo e siamo sicuri che tutti i cittadini beneficeranno di queste norme di grande buonsenso.

perché i dati che riguardano gli incidenti stradali e che descrivono il fenomeno di cui stiamo parlando sono purtroppo molto importanti e significativi. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei nostri giovani, dei ragazzi sotto i trent'anni, e secondo i dati del 2022 il tasso di mortalità stradale è pari a 53 cittadini ogni milione di abitanti, un numero nettamente più alto rispetto ai 26 morti del Regno Unito, ai 49 della Francia, ai 34 della Germania e ai 36 della Spagna: un dato che ci deve davvero far pensare e che dovrebbe spingerci a ragionare e non a fare battaglie ideologiche, come invece questo provvedimento intende fare intende fare (e fa). Il costo sociale degli incidenti stradali italiani ha toccato, nel 2022, 17,9 miliardi di euro ed è una cifra che corrisponde allo 0,94 per cento del PIL nazionale. Devo dire che non mi piace citare questo numero, perché le vite umane valgono enormemente di più; tuttavia è un numero, questo, che da chi governa e chi è chiamato a legiferare deve essere tenuto in considerazione. Voglio ricordare - è per questo che parlo di battaglia ideologica - che a Bologna, ragione per cui avete messo mano così velocemente a questo provvedimento, per contrastare fondamentalmente l'operato del sindaco di Bologna, nei pochi mesi di zona 30

e noi sappiamo che il numero più alto di morti per incidente stradale avviene in città e sono perlopiù pedoni. La Spagna, in un anno e mezzo, ha ridotto del 9 per cento i decessi sull'anno precedente.

perché c'era la campagna elettorale, e c'era l'illusione che la battaglia contro "velocità 30" della città di Bologna vi avrebbe portato voti; ma mi sembra che la risposta dei cittadini abbia parlato con molta chiarezza.

tra le scampanellate e i campanelli, la battaglia al 30, il racconto dei tombini, trovatene un'altra e provate a cambiare modo di fare politica nelle nostre città e nelle nostre zone perché, come vedete, i cittadini hanno la testa per capire di cosa si parla. Tornando alla questione di Bologna, che mi sta particolarmente a cuore, voglio ricordare che proprio due giorni fa, domenica 17 novembre, si è tenuto un presidio a Roma, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime sulla strada e che questa manifestazione, che non è certamente l'unica, si è accompagnata a un *flash mob* in diverse città italiane anche nei giorni successivi. E domani, quando si voterà il provvedimento, ci sarà un *flashmob* davanti al Senato contro la riforma del codice della strada voluta dal ministro Salvini,

o da grandi esperti, hanno definito una riforma di un Ministro forte con i deboli e debole con i forti. Essa infatti allenta le regole e i controlli per auto e camion, toglie spazi sicuri a pedoni e ciclisti, peggiora la sicurezza per tutti gli utenti della strada, attacca la mobilità sostenibile, togliendo autonomia alle città. città. Questi *flashmob* hanno luogo anche con riguardo alla legge di bilancio 2025 che taglia 154 milioni di investimenti su sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Ho ancora nelle orecchie le parole che Salvini urlava in campagna elettorale e ogni volta che lo abbiamo sentito parlare di questo argomento, quando poi, invece che prevenire gli incidenti, si lavora, come sempre, nel tentativo di aumentare i reati, crearne di nuovi, mettere sempre più gente possibilmente in galera, accompagnandoli magari con le parole che abbiamo sentito

Perseguirli ed essere severi con comportamenti inammissibili, come l'ubriachezza o altro, è assolutamente corretto, ma qui dobbiamo lavorare per la prevenzione e dentro questo provvedimento sulla sicurezza stradale sembra che questo non interessi.

ci troveremo con le associazioni italiane dei familiari delle vittime della strada, le associazioni ambientaliste e per la mobilità sostenibile e le organizzazioni sindacali a dare vita a un'altra nuova fase di mobilitazione che si svolgerà a Roma, ma non solo.

dimostra che c'è una profonda incapacità di ascoltare chi ha studiato e, purtroppo, come ho detto, ha vissuto anche il dramma di perdere un figlio giovane per un incidente stradale. legge è considerata in questo caso uno sfregio proprio perché è stata messa in coincidenza con la Giornata mondiale in memoria delle vittime. L'impianto di questa riforma è molto chiaro, perché dà maggiore libertà di circolare ai veicoli a motore, i cui guidatori, secondo i dati Istat, causano il 94 per cento degli incidenti e il 98 per cento dei morti; ed è forte, come ho detto, con i deboli perché restringe le misure in favore di pedoni, di ciclisti, di bambini e di persone anziane che sono la maggior parte delle vittime nelle città. È una riforma pericolosa perché limita gli autovelox invece che la velocità. [**Presidenza non so quanto possa premiarvi anche in termini di consenso, almeno a me non sembra, visti anche i risultati che la Lega, di cui il ministro Salvini è espressione, sta portando a casa. A me non pare che le persone stiano apprezzando questo tipo

che resta, come ho detto, la prima causa di collisione e di morte; vieta i controlli automatici sulla guida distratta al cellulare, che è - anche questa - tra i primi fattori di incidentalità; introduce una sola multa per più infrazioni, altra cosa di cui non capisco la *ratio*, anche come semplice cittadina non particolarmente esperta, se non appassionata di questo tema.

sbagliatissima nella sua filosofia ed è dannosa, perché rende più difficile creare o proteggere le aree pedonali, le piste e le corsie ciclabili, zone a traffico limitato e a basse emissioni, fondamentali per la tutela dell'incolumità e della salute delle persone nelle città. La riforma limita anche l'azione dei Comuni, sottoponendole a decreti ministeriali. Come ho detto, è stato evidente fin dal primo momento che c'è stata l'illusione che fosse un ottimo strumento di campagna elettorale, contro una città che, nella storia delle politiche della sinistra, è certamente una città emblematica, una città modello, vorrei dire. Naturalmente lo dico con l'umiltà di chi sa che non tutto è perfetto, ma certamente tutto si fa con il massimo dell'attenzione alla comunità, e tutelare una comunità significa tutelare, appunto, chi va protetto, in un momento in cui tutti sappiamo che le persone, i nostri giovani prendono sempre più volentieri la bicicletta per potersi muovere, perché è anche un elemento di salute.

dell'Organizzazione mondiale della sanità attesta che il numero di vittime della strada in tutto il mondo rimane inaccettabilmente elevato, con circa 1,35 milioni di morti ogni anno. Nell'Unione europea, tra il 2010 e il 2020, il numero di decessi dovuti a incidenti stradali è diminuito del 36 per cento, ossia una percentuale notevolmente inferiore all'obiettivo del 50 per cento stabilito dalla Commissione europea nel Libro bianco del 2011. Inoltre, l'obiettivo strategico degli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale di ridurre i decessi sulle strade del 50 per cento in quel decennio non è stato conseguito. Nel 2022 il numero delle vittime della strada - 20.640 persone - è di fatto aumentato del 4 per cento rispetto all'anno precedente. Pertanto, pur ritenendo significativo e cogente il proposito dell'Unione europea di dimezzare il numero di morti e feriti gravi sulle strade entro il 2030 e pressoché azzerarlo entro il 2050, bisogna obiettivamente ragionare sul fatto che con queste statistiche il numero delle vittime potrebbe diminuire entro il 2030 solo di un quarto, anziché della metà. Per raggiungere l'obiettivo intermedio sarebbe necessaria una riduzione annuale media del numero di decessi del 4 per cento, che però negli ultimi cinque anni è stata solo del 2,5 In Italia quest'anno fino al 10 novembre già contiamo un totale di 1.254 vittime; negli ultimi giorni ci sono stati altri 22 morti e solo ieri, nella Giornata mondiale in ricordo delle vittime degli incidenti stradali, cinque persone hanno perso la vita, tra cui due giovanissimi. Gli incidenti stradali rappresentano oggi la principale causa di morte tra i bambini e giovani adulti di età compresa fra i cinque e i ventinove anni e secondo quanto riferisce l'ONU costano alla maggior parte dei Paesi il 3 per cento del PIL, impattando perciò non solo sugli affetti, le vite e le famiglie, ma anche pesantemente sulle economie pubbliche. Roma e il Lazio, poi, sono purtroppo i detentori in Italia del triste primato per numero di vittime di incidenti stradali. È dunque un dovere morale e sociale, prima ancora che istituzionale, cercare soluzioni più efficaci e di lungo periodo per fermare questa strage. Concordo pertanto con il ministro Salvini quando dice che salvare vite è una missione che deve coinvolgere tutti ogni giorno, e anche sul fatto che chi non c'è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti. È significativo, perciò, portare in Aula il presente disegno di legge proprio durante questa settimana e riformare finalmente una legge elaborata nel 1959, quindi frutto di un tempo diverso, di socialità diverse e con tecnologie diverse. nuove tecnologie e nuove socialità rispetto a quelle degli anni Sessanta che, ad esempio, l'anno scorso hanno sconvolto la comunità di Acilia, dove io abito, quando un ventenne *youtuber* del canale collettivo «The borderline» alla guida di un bolide ad alta velocità ha ucciso il piccolo Manuel Proietti. Lo *youtuber* viaggiava a 100 chilometri orari su una strada il cui limite è di 50 e sotto effetto di marjuana. Da semplice cittadina desidero esprimere di nuovo la mia solidarietà ai familiari ancora sotto *choc* per quanto accaduto e al nostro quartiere colpito da una tragedia così grande, ma certamente evitabile. Come rappresentante delle istituzioni, invece, mi sento di dire che bisogna continuare a contrastare questo modello di cultura della trasgressione, che è sbagliato e che invoglia i giovani a vivere senza responsabilità, non facendoli rendere conto delle conseguenze che le loro azioni possono avere sulle vite umane, sui loro coetanei e forse anche sui loro amici e fratelli. Per questo era importantissimo intervenire con nuove regole per i neopatentati e per i minorenni che si mettono alla guida anche ubriachi e sotto effetto di droghe; era necessario, ancora, intervenire con multe più pesanti e controlli più severi per chi guida con il cellulare in mano e aumentare le sanzioni per eccesso di velocità; così come era importante incentivare le pene per chi si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e ad esempio di marijuana, ritenuta un bene da utilizzare a scopo ricreativo. A questo riguardo vorrei sottolineare quanto sia importante l'uso corretto delle parole. il rischio di inculcare l'idea che la cultura dello sballo sia una semplice ricreazione che non porta conseguenze, mentre non deve essere considerato un divertimento distruggere per sempre la vita e i sogni delle persone. Un recente studio dell'istituto americano per la sicurezza stradale, ad esempio, rileva che la percentuale di incidenti con lesioni e morti è aumentata nei mesi successivi all'allentamento delle leggi USA sulla marijuana: la legalizzazione nei cinque Stati avrebbe determinato un aumento del 6 per cento degli incidenti con lesioni e del 4 per cento di incidenti mortali rispetto agli Stati in cui era illegale. Sono dati che anche l'Italia deve prendere considerazione; ben venga, perciò, la revoca della patente se l'automobilista risulta positivo ai test salivari. La prima forma di prevenzione, però, prima ancora del sanzionare efficacemente questi comportamenti, per non avere più morti in strada è promuovere la cultura della vita e del vivere sano, al contrario di quanto fa troppe volte la sinistra, soccombendo al fascino di deresponsabilizzare l'uso della *cannabis* e affini. La formazione deve iniziare fin dalla giovane età, per inculcare nei nostri ragazzi una cultura della sicurezza che li accompagni per tutta la vita. Investire nell'educazione, nella consapevolezza e nella cultura della sicurezza è fondamentale per proteggere le vite e garantire un futuro migliore per le generazioni. Per questo è doveroso. Ho letto poi anche di qualche strumentale polemica, ma per concludere desidero ringraziare non solo il Governo, ma anche tutte le associazioni che, indefessamente, da decenni si battono per la tutela delle vittime e dei loro familiari. È vero che con molti di loro abbiamo collaborato in questi anni, avendo pure qualche divergenza di vedute, la certezza che lo spirito ultimo deve essere - e questo è - evitare tragedie che sconvolgono le famiglie e che non devono avere alcuna giustificazione. Vorrei salutare da questo banco l'avvocato Cesari, ormai non più fra noi, esempio straordinario di impegno in questo campo, missione portata avanti con determinazione proprio dopo essere stato investito lui stesso trent'anni fa sulle strisce pedonali. Vorrei anche ringraziare Pina Cassaniti Mastrojeni, esemplare modello di madre coraggio che, dopo quella sera d'estate del 1997 che le portò via la figlia, ha dedicato la sua vita, con impegno, passione, costanza e ammirevole ostinazione, alla tutela dei diritti e della giustizia per le vittime della strada. Desidero quindi rassicurare che il loro obiettivo è il nostro ed è quello di creare un quadro normativo che funzioni da forza deterrente affinché si fermino le stragi sulle strade. bisogna chiarire una volta per tutte che la mobilità dolce non è sempre la risposta adatta ed esaustiva alla prevenzione dell'incidentalità. Le zone 30 non sono la panacea di tutti i mali. Bisogna avere il coraggio di dirlo. In primo luogo, le zone 30 sono zone, dunque porzioni di territorio comunale, non interi Comuni. Le zone 30 sono nate, infatti, con una logica specifica, cioè quella di elevare l'attenzione in determinati punti della città, come le scuole e gli asili, dove è importante e soprattutto utile sollecitare un passo allentato delle auto. Di contro, forzare la percezione degli automobilisti e dei cittadini, obbligandoli con ordinanze amministrative a viaggiare a bassissima velocità, risulta una direttiva poco applicabile, ma anche deleteria, perché di fatto produce più inquinamento, triplica i tempi di percorrenza per andare al lavoro o semplicemente per spostarsi e adduce un danno ai tessuti produttivi. Ricordo, infine, che la prima causa di incidentalità stradale è la distrazione. Distrazione che può aumentare proprio durante una guida più calma. Bene ha fatto, pertanto, il Ministero a fermare questo furore ideologico, questa nuova moda di mettere la bandiera sulla sicurezza stradale, facilmente smontata anche da alcune statistiche che ricordano, ad esempio, che la maggior parte degli incidenti con feriti gravi e mortali avviene in ambito extraurbano e non nei Comuni. Fermiamo subito tutte quelle scelte che, in nome di una paventata sicurezza, vorrebbero imporci un nuovo confinamento. Non facciamo l'errore di creare un *lockdown* delle auto, ma ragioniamo. Infine arriviamo a loro, ai monopattini elettrici, che finalmente dovranno avere assicurazione, targa e freccia obbligatoria. Finalmente sarà obbligatorio l'uso del casco, sarà vietato parcheggiarli casualmente sui marciapiedi, non potranno più circolare fuori dai centri urbani, sulle strade extraurbane ed in galleria. Era davvero giunta l'ora di mettere ordine, oltre che per una questione di sicurezza, anche per l'occupazione incontrollata del suolo pubblico, per contrastare gli atti di vandalismo, cui abbiamo assistito anche nella Capitale con il lancio dei monopattini nel fiume Tevere. Avanti così, dunque, con queste nuove regole e con tutte le scelte che, senza pregiudizi e con molto buonsenso, ci vedono determinati a rendere le nostre strade più sicure, a ridurre gli incidenti; e che queste regole ci aiutino a raggiungere seriamente l'obiettivo di arrivare a zero morti.

3.039 e 1.254. Il primo numero rappresenta le vittime di incidenti stradali in Italia nel 2023. Il secondo indica i morti sulle nostre strade dall'inizio dell'anno fino a una settimana fa. Questo significa che, ogni mese, abbiamo visto 114 vittime, il che si traduce in quattro persone che perdono la vita ogni giorno. È come se quotidianamente perdessimo una famiglia intera. Questi numeri nascondono storie drammatiche: famiglie distrutte da un attimo di distrazione, da una curva pericolosa o da una serata di eccessi. Con questo disegno di legge stiamo avviando una profonda revisione del codice della strada, che attendiamo da oltre trent'anni. Un tagliando necessario, che risponde a un contesto ormai in continua evoluzione. La micromobilità, per esempio, con la diffusione di monopattini elettrici e biciclette assistite, ha aggiunto una nuova dimensione al dibattito sulla sicurezza stradale, contribuendo ad un incremento preoccupante degli incidenti, spesso coinvolgendo i nostri ragazzi. Finalmente introdurremo l'obbligo del casco per monopattini. Se fosse per me, renderei obbligatorio per tutti i monocicli addirittura il casco integrale, che dimezza la probabilità di subire lesioni al volto, dimezza la gravità dei danni permanenti. E se metà di quest'Assemblea avesse visto, in pronto soccorso, da incidenti in motorino, anche urbani, sono certa che la penserebbe come me. Quindi, bene il casco per i monopattini. Parliamo sempre di sicurezza e non può prevalere solo la logica della salvaguardia delle aziende. La vita vale più del fatturato delle società di noleggio dei monopattini. *(Applausi)*. Non possiamo più ignorare le nuove cause di incidenti. Dopo la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, oggi miete vittime la distrazione alla guida causata dall'uso del telefonino: inviare messaggi su WhatsApp riduce i tempi di reazione al volante come quattro birre medie. Scattarsi un *selfie* o pubblicare una storia sui *social* richiede almeno secondi di distrazione; accedere a un *social* per scoprire quanti *like* abbiamo guadagnato significa distrarsi per venti secondi; chi invia un messaggio alla guida distoglie gli occhi dalla strada per circa 4,6 secondi. Questo, a una velocità media di 50 chilometri all'ora, equivale a percorrere la lunghezza di un campo da calcio a occhi bendati. I tempi di reazione, in caso di possibile impatto, si riducono quindi del 35 per cento. Da oggi chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare mentre guida dovrà affrontare sanzioni severe, con il ritiro della patente da quindici giorni a due mesi, e multe che possono arrivare a 1.600 euro. In caso di recidiva, le conseguenze saranno ancora più gravi. Ventidue anni fa ho fatto un incidente che ha avuto quasi del miracoloso perché, proprio per rispondere al telefono, non diedi la precedenza a una macchina e per evitarla

ancora più necessaria oggi per mettere in guardia chi vive la guida come un'avventura superficiale e per garantire la sicurezza di tutti. Infatti, la guida non è un gioco e nessuno può permettersi di mettere a rischio la vita degli altri. Le nuove disposizioni non si fermano qui. Per la prima volta l'omicidio stradale viene riconosciuto riconosciuto come un reato grave, con pene che prevedono fino a dieci anni di sospensione della patente e che possono arrivare a trent'anni in caso di recidiva. È fondamentale che chi causa danni irreparabili alla vita di un altro venga chiamato a rispondere delle proprie azioni. Siamo anche determinati a garantire un accertamento rigoroso delle violazioni utilizzando tecnologie avanzate come telecamere e dispositivi di controllo, un modo per tutelare la sicurezza di pedoni e ciclisti e per sanzionare comportamenti irresponsabili. Inoltre, per garantire la sicurezza dei cittadini i neopatentati potranno guidare solo auto di media cilindrata. È una legge della fisica: più si va veloci e più aumentano i tempi di reazione a un evento e di frenata per evitarlo.

per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati alle infrazioni stradali. È fondamentale che i nostri giovani comprendano che guidare in sicurezza e rispettare le regole è un beneficio prima di tutto per loro e, poi, anche per gli altri. In conclusione, il codice della strada che approviamo oggi rappresenta la nostra visione basata su pragmatismo, sicurezza e tutela dei cittadini, senza favorire l'anarchia in nome di un'ideologia cieca che costringe i cittadini a muoversi solo con i monopattini o mezzi elettrici, seguendo direttive di qualche burocrate di Bruxelles, senza installare *autovelox* a ogni angolo della strada per fare cassa (noi riteniamo che i limiti di velocità debbano essere rispettati con criteri uniformi in tutto il Paese), senza trasformare le ZTL in una sorta di girone dantesco per cui chi entra accidentalmente in una zona vietata viene punito con sanzioni multiple, e prevedendo regole affinché le piste ciclabili siano sicure e non solo degli *spot* elettorali

nonostante tanti proclami e forzature, in decenni di potere la sinistra non ha mai modificato l'impianto normativo. Oggi sono in vigore norme stabilite con un decreto del 1992: parliamo di oltre trent'anni fa, quando la gente si muoveva in tutt'altro modo e il piano urbanistico era decisamente più elementare. Questo Governo e il ministro Salvini, che ringrazio, hanno avuto il coraggio di mettere seriamente mano al codice della strada con un provvedimento fondamentale atteso da decenni, il cui obiettivo primario è ridurre gli incidenti e le vittime sulle nostre strade. è stato anche portato avanti attraverso il dialogo con esperti, con i cittadini, attraverso una consultazione pubblica promossa dal Ministero delle infrastrutture, che ha permesso di raccogliere idee e proposte per un codice efficace e anche attuale. Abbiamo bisogno quindi di un equilibrio tra prescrizioni e sanzioni, perché la nostra priorità priorità deve essere quella di tutelare chi rispetta le regole. Lavoriamo insieme per un futuro più sicuro per tutti, certi che i cittadini saranno dalla nostra parte.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti di Governo, desidero iniziare il mio intervento sul provvedimento oggi in discussione qui in Aula, il codice della strada, andando subito al nocciolo della questione e leggendo quanto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini ha postato tre giorni fa, in occasione della Giornata mondiale delle vittime sulla strada. Esordendo con il titolo «In omaggio alle vittime arriva nuovo codice», Salvini, scrive: «la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada anticipa di pochi giorni l'approvazione del nuovo codice, che ho voluto fortemente dopo decenni di attesa e dopo troppe tragedie, che troppo spesso coinvolgono ragazze e ragazzi. Siamo determinati a rendere le nostre strade più sicure, riducendo gli incidenti che spesso sono figli di distrazione imprudenza. Nell'ultimo anno abbiamo ascoltato anche associazioni, enti locali, produttori automobilistici, esperti. Salvare vite è una missione che deve coinvolgere tutti, ogni giorno, oltre ogni schieramento politico. Chi non c'è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti». Questo è quello che ha scritto il ministro Salvini. Sembra troppo bello per essere vero, troppo umano, troppo nobile, quello che scrive il Ministro. Infatti vero non è, tanto che oggi desidero leggervi alcune righe di una lettera che mi è stata inviata da Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, famoso ciclista su strada che vinse anche il Giro d'Italia del 2011, morto in un incidente stradale, investito da un furgone mentre si stava allenando sulle sue strade.

i miei genitori, mia sorella, non hanno scelto di diventare quello che sono oggi. La tragedia che ci ha colpito sette anni fa con la morte di Michele ci ha portato a reagire impegnandoci ogni giorno per una nuova strada che salvaguardi più vite umane possibili. Noi e tanti come noi abbiamo creato associazioni, fondazioni; entriamo nelle scuole, promuoviamo occasioni di confronto, incontriamo cittadine e cittadini ogni giorno. Alcuni di noi sono diventati veri e propri tecnici della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Se qualcosa è cambiato in meglio in merito a questi aspetti nel nostro Paese, lo dobbiamo anche a loro. Abbiamo aspettato tanto tempo, troppo, che il codice della strada, quel patto stretto tra noi per condividere la strada in pace, cambiasse mettendo al centro finalmente una visione giusta, nuova, con la persona e la vita al primo posto e con tutte quelle riforme necessarie per favorire una vera cultura della sicurezza stradale e della mobilità attiva e sostenibile. Confidavamo davvero che queste modifiche fossero una risposta a un passato e a un presente ancora di dolore e ci aprissero a un futuro di speranza. Purtroppo non è così. Non è corretto che il Governo dica che ha ascoltato le associazioni di familiari delle vittime. *(Applausi)*. Le ha fatte parlare, ma non le ha ascoltate non ha preso niente di quanto è stato detto nelle audizioni. Queste sono le parole di Marco Scarponi. E in un *post* la Fondazione Scarponi, nella Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, riferendosi al nuovo codice della strada, aggiunge: fa ancora più male che queste scelte vengano giustificate facendo continuamente riferimento alle vittime della strada e alle loro famiglie. Questo atteggiamento non solo tradisce le aspettative di chi crede in una mobilità più sicura, ma ferisce profondamente coloro che hanno già pagato un prezzo altissimo. Oltre alla Fondazione Scarponi, tantissime per non dire tutte le associazioni dei familiari delle vittime della strada contestano la tremenda e disumana strumentalizzazione fatta dal ministro Salvini sulle spalle di chi oggi non ha più voce, perché vittima di un incidente stradale, ma fatta anche sulle spalle di intere famiglie straziate da lutti dovuti a questi incidenti, famiglie che in un istante hanno perso persone amate, amiche e amici, giovani bambine e bambini. Ritengo che sia nostro dovere morale dare voce a queste associazioni e parlare di fatti concreti e del mondo reale, non del mondo fittizio creato *ad hoc* senza vergogna di chi ha voluto questo codice della strada non di certo per aumentare la sicurezza stradale, ma per altri interessi, palesati fra l'altro nello stesso *post* di Salvini, quando menziona solo i produttori automobilistici, dimenticandosi di tutti gli altri produttori Aurora). Queste associazioni - come è stato detto prima anche dalla collega Zampa - in un comunicato hanno messo nero su bianco la loro contrarietà. Non potete continuare a dire che state approvando un provvedimento per omaggiare le vittime della strada. Non potete dirlo.

peggiora la sicurezza per tutti gli utenti della strada, attacca la mobilità sostenibile. Abbiamo sentito adesso parlare la collega Ronzulli, ma anche la collega Pellegrino, attaccando la mobilità sostenibile. Diciamoci la verità, almeno qui nell'Aula del Senato: il codice della strada oggi in discussione, soprannominato "codice della strage" proprio dalle associazioni che si occupano e si preoccupano di sicurezza stradale, è stato scritto in barba alle raccomandazioni e alle richieste che tutte le più importanti associazioni dei familiari delle vittime hanno presentato unite più volte. Nessuna loro richiesta è stata accolta: zero. Quindi le associazioni sono state barbaramente strumentalizzate. Stasera Stasera mi sarei augurata, colleghe e colleghi della maggioranza, che almeno in quest'Aula non avreste avuto il coraggio di offendere di nuovo la dignità di chi ha perso persone care in incidenti stradali. Evitate, per favore, per rispetto loro, di omaggiare chi ha perso la vita in incidenti stradali, volendo farci credere che il nuovo codice della strada salverà vite. Abbiate invece il coraggio di spiegarci bene la vera visione antiquata che avete della circolazione e della sicurezza futura sulle strade italiane, perché purtroppo, per come è stato scritto il nuovo codice della strada, la sicurezza stradale rimarrà un miraggio. Dovremo continuare a percorrere, anche in futuro, strade piene di pericoli, con pedoni e ciclisti considerati come birilli fastidiosi che intralciano la circolazione delle macchine, e continuare ad accettare che siano le auto le padrone delle nostre città, periferie, territori e anche località turistiche, costringendoci a un percorso ad ostacoli, rendendo più difficile il movimento in sicurezza di tutte le persone, anche sugli stessi marciapiedi. Penso alle fasce più fragili, alle persone anziane, alle mamme con carrozzine, alle persone con disabilità, alle bambine e ai bambini che i genitori italiani non fanno più andare a scuola a piedi perché terrorizzati dalla giungla stradale. Dobbiamo quindi rassegnarci? La vita non è uno scherzo, così inizia una poesia di Nazim Hikmet. Va presa sul serio, ancora più sul serio da chi, come noi in quest'Aula, ha la possibilità concreta di salvare vite e ha una responsabilità istituzionale nei confronti Come persona che ha vissuto sulla propria pelle la perdita di tante persone care, vittime di incidenti stradali, convinta che qui in Aula ognuno di noi abbia una lista riservata di persone altrettanto care che avrebbero potuto e voluto essere ancora qui tra noi oggi, dico, anche a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, che non ci rassegniamo al voto finale al Senato, che teoricamente e umanamente, colleghe e colleghi della maggioranza, potreste ancora influenzare. Da parte nostra appoggeremo la mobilitazione futura delle associazioni, già annunciata questi giorni, ringraziandole di cuore per il loro preziosissimo lavoro quotidiano, volto a promuovere una vera cultura ed educazione alla sicurezza stradale, che questa maggioranza non ha ritenuto voler contemplare nel nuovo codice della strada. La vita non è uno scherzo, prendiamola e prendetela sul serio.

i miei colleghi di Commissione lo sanno. Intanto vorrei precisare, perché raccolgo diversi pensieri su questo che la necessità dell'intervento normativo è stata ravvisata in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli estremamente elevati di incidentalità: nel 2023 sono 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia, 224.000 i feriti, 166.000 gli incidenti stradali. I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, in leggera diminuzione per le vittime, che rimangono però elevatissime. che otto persone al giorno muoiano ancora sulla strada, nonostante i passi avanti che sono stati fatti in tema di sicurezza, è preoccupante e merita nuove norme più restrittive. Le vittime aumentano nel 2023 anche per i conducenti di monopattini, di biciclette e di biciclette elettriche. Per le biciclette e le biciclette elettriche siamo purtroppo a 212 vittime,

Se guardiamo all'Unione europea, ogni milione di abitanti si contano 45 morti per incidente stradale, mentre nel nostro Paese

Infine, su un totale di 52.459 incidenti con lesioni, osservati da Carabinieri e Polizia stradale, sono più di 5.000 quelli con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di ebbrezza e 1.700 quelli per i quali si è rilevato l'effetto di stupefacenti. Nel complesso, sono dati molto preoccupanti. Ecco perché il disegno di legge vuole dare risposte a tali preoccupazioni con con un ampio pacchetto di modifiche che ruota anzitutto attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, che include anche modifiche al codice penale su omicidio stradale e lesioni stradali, volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada, in particolare eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psicofisica. Sempre con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa, viene rivisitato il sistema della patente a punti. Infatti, nel nuovo regime, dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti, non segue più soltanto l'ulteriore decurtazione del punteggio, ma viene irrogata anche la sanzione della sospensione breve della patente. La riforma proposta poi interessa gli aspetti della formazione dei guidatori, della gradualità dell'abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e dell'accertamento della violazione con strumenti da remoto. remoto. Il testo proposto concerne inoltre le tematiche dei veicoli di micromobilità elettrica e della circolazione delle biciclette, con modifiche volte a migliorarne la sicurezza. A chiusura del provvedimento, il disegno di legge comprende un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all'autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione. Sono stati numerosi, nel corso dell'esame alla Camera, gli emendamenti di Forza Italia approvati. Anche al Senato, dopo una serie di audizioni, abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti volto a migliorare ulteriormente il testo nella direzione della sicurezza e della prevenzione. In considerazione però dell'urgenza dell'entrata in vigore di queste norme, che prevedono molte disposizioni salvavita, abbiamo convenuto che un nuovo passaggio alla Camera ne avrebbe rinviato troppo a lungo l'applicazione. Abbiamo quindi ritenuto di convertire gli emendamenti più significativi in ordini del giorno vincolanti.

Abbiamo quindi impegnato il Governo a rivedere la disciplina speciale relativa ai neopatentati, intervenendo sulle ipotesi di limitazione alla guida in rapporto a un determinato periodo di tempo e in relazione ai limiti di potenza. Se è giusto portare da un anno a tre anni il periodo in cui i neopatentati hanno limitazioni in termini di potenza delle vetture guidate, non ci sembra coerente l'aumento, seppur minimo, della potenza stessa rispetto alla norma attualmente vigente. Abbiamo impegnato il Governo a fornire indicazioni precise in merito alla necessità di assicurare concreta attuazione a quanto previsto in relazione ai contenuti della prova teorica, riferiti alle fattispecie che generano maggiore incidentalità, inserire cioè l'insegnamento a scuola guida degli effetti di alcol e droga, di elementi di primo soccorso, spiegare quali sono i fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada, in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio giorno-notte e dei fattori di rischio specificatamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada. Abbiamo impegnato il Governo a rivedere e definire, ferme restando le vigenti attribuzioni degli organi di polizia nell'espletamento dei servizi di polizia stradale, il novero degli ulteriori soggetti abilitati all'espletamento delle funzioni di polizia stradale e relativi ambiti di competenza. Troppe volte i Comuni utilizzano personale non qualificato per servizi di polizia stradale. Grazie a questo ordine del giorno il Governo metterà ordine. Abbiamo parlato anche di rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate per le violazioni del codice della strada, chiarendo in particolare da quali soggetti saranno incassate le stesse e quale dovrà essere la destinazione dei relativi proventi, assicurando la destinazione prioritaria a interventi di riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale, oltre che alla manutenzione delle strade e al costante aggiornamento della segnaletica. Purtroppo non tutti gli enti locali utilizzano i proventi delle multe per aumentare la sicurezza stradale. Noi vogliamo invece che sia così. Vogliamo che i soldi di chi viola il codice servano per rendere più sicure le strade, per salvare le vite e non per tappare buchi di bilancio. Ecco perché abbiamo impegnato il Governo anche a monitorare le rendicontazioni effettuate dagli enti locali.

quella che c'è sul retro, anche in capo ai veicoli di vecchia immatricolazione e in particolare ai mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone, i pullman. Pensate che, una volta tanto, siamo stati copiati dall'Europa, perché la norma della segnalazione della sagoma dei TIR è entrata in vigore in Italia e poi l'Europa ci ha copiato. Con questo ordine del giorno impegniamo il Governo a far sì che lo faccia anche sui pullman, che tra l'altro non trasportano merci, ma trasportano persone e, quindi, è ancora più importante. Abbiamo impegnato il Governo anche a rivedere in modo organico la disciplina sui limiti di velocità, rivalutando eventualmente l'inasprimento delle sanzioni alla luce di un'attività di monitoraggio. Abbiamo rilevato che l'articolo 35 del disegno di legge collega la dissuasività della sanzione anche alla situazione reddituale del soggetto, la multa si paga in base alla dichiarazione dei redditi. Abbiamo voluto specificare che, in sede di attuazione della delega, questo principio venga interpretato non nel senso di alzare le sanzioni a chi ha un reddito più elevato, mantenendole immutate per i meno abbienti, ma invece di ridurre l'importo delle sanzioni per i meno abbienti, mantenendo inalterate le altre. dovrà, inoltre, promuovere in via amministrativa, a seguito del completamento della sperimentazione del progetto IT Wallet e della patente digitale, meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida con modalità semplici per l'utente. Lo Stato deve essere amico del cittadino: se impone il rinnovo di un documento a lunga scadenza, è giusto che almeno avvisi il cittadino della prossima scadenza dello stesso. Dovrà prevedere un importo massimo da corrispondere determinato in misura proporzionale, sulla base della categoria del veicolo, del tipo di emissione, della classe, nella delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL da parte dei Comuni: norma necessaria per uniformare, almeno nell'importo massimo, i costi delle ZTL, che in Italia a volte sono eccessivi. Come sapete qui in Senato e in Parlamento abbiamo modificato la Costituzione per inserirvi lo sport. Ebbene, viene naturale modificare in tal senso anche il codice della strada, prevedendo che sulle strade e aree pubbliche siano permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, ribaltando la vigente normativa, che prevede che le competizioni sportive su strada siano vietate, salvo delibera che le autorizzi. La vigente normativa dissuade il cittadino dal fare opposizione a una sanzione di scarsa entità, in quanto il contributo da versare a volte è maggiore della sanzione stessa. Dobbiamo permettere al cittadino di difendersi da eventuali errori commessi nell'irrogare la sanzione. Ecco perché abbiamo impegnato il Governo ad adottare disposizioni volte a individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo unificato e comunque la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell'opposizione. Purtroppo è in aumento il numero delle persone che non provvedono a versare l'importo delle sanzioni, obbligando i Comuni a costose e impegnative operazioni di recupero crediti che non sempre vanno a buon fine, anzi. Ecco perché abbiamo proposto di individuare meccanismi effettivamente premiali, che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti, decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione più alta, rispetto all'attuale, dell'importo della sanzione prevista. Tale disposizione aiuterebbe i comuni a rincorrere di meno i trasgressori e avere entrate più certe. Per quanto riguarda la micromobilità, abbiamo lavorato per rendere le norme più eque. Intanto - come sappiamo tutti - un monopattino non è un'autovettura e per abbiamo impegnato il Governo a tener conto delle diverse esigenze che ricorrono in materia di assicurazione dei monopattini, al fine di assicurare che la stessa risulti proporzionata, in termini di onerosità, ai potenziali effetti lesivi del dispositivo, che sono inferiori rispetto a quelli conseguenti dai veicoli a potenza e cilindrata superiore. È evidente che i danni che possono provocare un monopattino o una bicicletta sono inferiori a quelli che al problema del casco, di cui ha parlato anche la collega, presidente Ronzulli. Devo dire che mi ha stupito la norma che prevede l'obbligo del casco per i monopattini elettrici, mentre

Tre anni fa, quando tutti insieme eravamo alla Camera - c'era il Governo Draghi - elaborammo l'ultima proposta sulla micromobilità che divenne legge; in quella sede

Nel 2023 i morti che guidavano una bicicletta sono stati 212, mentre i morti utenti del monopattino sono stati 21.

il monopattino in città; mentre mia figlia di undici anni, che ancora non conosce bene tutte le regole, può guidare di notte senza casco o su una strada provinciale. Questo è evidentemente uno dei problemi che abbiamo sottoposto al Governo,

a perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e della prevenzione degli incidenti stradali, con particolare riguardo all'uso di sistemi personali (quindi dei caschi), da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi, nell'ottica di una disciplina organica che possa configurare nel codice regole certe e proporzionate. Si tratta, quindi, di un'apertura all'inserimento del casco anche per chi va in bicicletta. un altro ordine del giorno propone di adottare regole chiare in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi, nonché misure per la tutela dei ciclisti e dei conducenti di velocipedi, tenuto conto delle relative caratteristiche tecniche. Infine, su questa materia abbiamo rilevato che, se è pur giusto salvaguardare la vita e l'incolumità della persona che guida il monopattino, quindi costringerla a mettere il casco, ciò ha una ricaduta negativa sullo *sharing* - questo è evidente per tutti - che ha circa 5.000 dipendenti in Italia e che evidentemente rischia, se non di chiudere, di essere molto ridotto. Abbiamo impegnato il Governo a valutare l'impatto della misura sui posti di lavoro delle aziende di *sharing*, immaginando soluzioni volte a conciliare la tutela della sicurezza stradale e l'uso del casco con le specifiche caratteristiche ed esigenze del comparto. Peraltro, questa norma entra in vigore immediatamente, forse sarebbe stato meglio dare qualche mese per adeguarsi. E, quindi, può essere un suggerimento per il Governo quello di dare anche una mano a queste aziende a non chiudere, mantenendo però la sicurezza con il casco obbligatorio. In sintesi, sono soddisfatto sia del fatto che anche il Senato abbia potuto approfondire tematiche che interessano la vita quotidiana di tutti gli italiani, sia che il Governo abbia riconosciuto la validità delle nostre proposte e delle osservazioni che gli abbiamo sottoposto. dicendo che fa male pensare che durante il tempo di questo dibattito, secondo le statistiche, in Italia una persona è morta sulla strada. Sono però convinto che abbiamo lavorato duramente per migliorare la sicurezza di tutti e per ridurre quei lutti improvvisi e strazianti che ancora troppe famiglie provano tutti i giorni.

per il suo tramite mi rivolgo al senatore Rosso, ringraziandolo per aver condiviso con quest'Aula il testo aggiornato di questo

l'attività del senatore Rosso è stata quella che avrebbe, in realtà, dovuto svolgere l'Aula, secondo i canoni e quindi con un ulteriore passaggio. Questo perché stiamo parlando non di una leggina, ma del codice della strada. Stiamo parlando di una legge che regolamenta il comportamento sulla strada di tutti i cittadini. Sinceramente, mi pare che meritasse di essere affrontata con la maggiore attenzione possibile e, quindi, eventualmente, anche con un ulteriore passaggio tra Camera e Senato. Come possiamo verificare dai venti minuti di descrizione del senatore Rosso,

dell'*iter* bizzarro e anomalo che sta seguendo l'approvazione di questo provvedimento che, viceversa, meritava ben altra attenzione secondo i canoni istituzionalmente previsti. Quindi, bene questa riforma, perché dopo più di trent'anni sicuramente il mondo è cambiato e la mobilità è cambiata. Abbiamo la consapevolezza che la visione auto centrica sia da abbandonare a favore del trasporto collettivo, del trasporto pubblico locale e della mobilità dolce; anche perché, con la situazione di inquinamento nelle più grosse città, lo favorisce. Questo, però, è il mondo dei sogni e il ministro Salvini evidentemente ha sogni diversi, sogni controcorrente o meglio, in questa circostanza, sogni contromano. Sappiamo tutti che la circolazione stradale causa ogni anno migliaia di morti e sappiamo tutti che le vittime della strada

È stato considerato che, nel primo semestre del 2024, sono aumentati dell'8 per cento gli incidenti nelle aree urbane rispetto al semestre scorso. Questo è un tema sensibile, a cui tutti fanno riferimento, perché come si fa a non essere sensibili allo stravolgimento che avviene nella vita di una di una famiglia che perde un caro a causa della sua morte in un incidente stradale? Infatti viene ricordato come *"that day"*, il giorno in cui tutto è cambiato. Quindi, anche le forze di maggioranza non fanno a meno di appellarsi a questi drammi. Nello stesso tempo, per esempio, visto che gli incidenti si verificano in zone urbane, per quanto riguarda la zona 30, vanno a limitare l'autonomia del Comune. Ma chi meglio di un sindaco conosce le aree pericolose che necessitano, in ogni caso, un intervento di questo genere? La casistica dice che, quando vengono introdotte le zone 30,

città o che riconosce come critica, il restringimento della carreggiata e la creazione di musoni. Dove ci sono gli attraversamenti pedonali sporgono due piccole isole in modo che il conducente, quando arriva, vede i pedoni già quasi al centro della strada e si arresta. Penso anche all'evidenziazione delle strisce pedonali con un leggero rialzo e magari fatte di un colore diverso, oppure a una strettoia o a una *chicane*. Ci sono esperienze europee molto diffuse.

altro punto critico è che sono stati tagliati i fondi per agevolare il trasporto pubblico locale. E c'è poi la grossa questione del cumulo delle sanzioni. sanzioni. Si prevede che, se nell'arco della stessa giornata, nell'ambito dello stesso ente pubblico - immaginiamo un Comune - venga comminata più di una sanzione, verrà applicata una sola sanzione: la più grave aumentata di di un terzo. Provo a immaginare il superamento del limite di velocità in città. Il superamento del limite può essere da 10 a 40 chilometri

alcuna colpa, se non quella di essere capitate nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è poi il tema dei neopatentati. Mi chiedo davvero per quale ragione bisogna aumentare la cilindrata dei veicoli che possono guidare. Le principali ragioni degli incidenti sono la velocità, la distrazione e la precedenza. Stiamo parlando di guidatori inesperti, che magari non sanno bene come muoversi sulla strada

aggiungiamo pure la velocità perché, se aumenti la cilindrata, aumenti anche il potenziale di velocità della macchina. Se poi aggiunge anche il testosterone, abbiamo fatto veramente tombola. Perché diamine vogliamo aumentare la cilindrata delle auto che mettiamo in mano ai nostri ragazzi? Non leggiamo le cronache, non vediamo che cosa succede al rientro dalle discoteche? Forse perché si usa la macchina del papà e allora non si può costringere il papà ad avere una cilindrata inferiore. C'è però anche lo *sharing*; ci sono altri modi per risolvere questa situazione. Si tratta quindi di una norma importante, ma viene trattata con superficialità fretta - la supervelocità causata dalla fretta - e poteva essere fatta meglio. Voglio solo sottolineare che ho presentato due altri emendamenti sui corridoi faunistici: una cosa fondamentale. Se non prevediamo i passaggi per la fauna selvatica, in modo che possano allargare il proprio spazio in altre aree, creiamo incidenti stradali, perché gli animali proveranno lo stesso ad attraversare le strade. E creiamo problemi anche a zone come il Trentino, dove per esempio gli orsi potrebbero portarsi nelle aree più interne, ma non possono farlo perché ci sono le barriere stradali. Se non gli facciamo i corridoi,

quando ormai veramente è una visione non degna di un Paese civile. Ho quindi presentato un emendamento anche in questo senso. Se il Governo vorrà creare tre ordini del giorno vincolanti, come le proposte da me presentate, aspetterò di vedere gli esiti.

nel 2023 i morti in incidenti stradali in Italia sono stati 3.039, 224.634 i feriti e 166.525 gli incidenti stradali. Secondo stime preliminari riportate in occasione della Giornata internazionale per le vittime della strada (17 novembre), nel semestre gennaio-giugno del 2024 si è registrato, rispetto allo stesso periodo del 2023, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (80.000, più quasi l'un per cento), dei feriti (107.643) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.429, più 4 dati che - lo dico a questa Assemblea - fotografano una situazione drammatica del nostro Paese. Per questo motivo, il lavoro del ministro Matteo Salvini per invertire la rotta deve essere condiviso, sostenuto e applaudito. Lo Stato non può rimanere inerme di fronte alle continue stragi stradali, e finalmente con questo disegno di legge si aggiornano delle misure ormai obsolete al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Tra le principali misure adottate nel provvedimento in esame vi è il rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol, con l'introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti, soprattutto quelli già condannati per reati specifici; nonché l'obbligo per gli stessi di installare i cosiddetti alcolock, ossia il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Sarà inoltre punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psicofisica, guidare avendo assunto droghe, con una modifica molto importante: ad oggi, incredibilmente, se un agente della Polizia stradale ferma una persona e questa risulta positiva al droga test, è onere dell'agente di pubblica sicurezza dimostrare che quella persona è in stato di alterazione. Con le nuove norme, invece, sarà punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psicofisica, guidare avendo assunto droghe. E la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e successivamente anche il divieto di conseguire il titolo di guida per ben tre anni. Il messaggio è chiaro: se ti droghi, non puoi guidare. Altro intervento riguarda l'uso del cellulare, una misura più che mai necessaria, perché almeno un quarto degli incidenti stradali con morti e feriti è causato dall'uso scorretto dello *smartphone* mentre si guida. Stando ai dati resi noti lo scorso mese di ottobre, è emerso che il 10 per cento degli italiani utilizza il dispositivo mobile per registrare video mentre guida. Gli automobilisti sorpresi con lo *smartphone* in mano durante la guida, e che abbiano almeno 10 punti sulla patente, subiranno una sospensione della stessa per sette giorni. La durata aumenta a quindici giorni se i punti residui sulla patente sono chiaramente meno di 10 e i tempi di sospensione raddoppiano in caso di incidenti causati dall'uso del cellulare. Per quanto riguarda i neopatentati, su cui abbiamo sentito prima alcune indicazioni da parte fermo restando il divieto per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guidare veicoli ad alte prestazioni, al fine di tener conto di un'esigenza importante delle famiglie con difficoltà economiche, costrette ad acquistare un'auto per i figli perché il limite dei kilowatt disponibili era molto basso, lo abbiamo innalzato prevedendo una potenza specifica di circa 130 cavalli. Non si tratta comunque di auto ad altissime prestazioni: questo limite dà la possibilità alle famiglie di dare ai propri figli la macchina, che magari è già di loro proprietà, evitando di gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini italiani. Per quanto riguarda l'autovelox - ho sentito delle critiche in precedenza su questo provvedimento - basta con l'anarchia degli impianti ovunque. Gli autovelox non devono servire per fare cassa, ma devono essere strumenti di assoluta prevenzione. Si prevede quindi di omogeneizzare la strumentazione utilizzata sul territorio nazionale, consentendo l'uso di apparecchi che siano approvati dal Ministero, predisponendo così un sistema unico, riconosciuto ugualmente in tutta Italia, che verrà ulteriormente rafforzato grazie al decreto interministeriale, con il quale saranno omologati i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocità uniformemente in tutta Italia. questa misura importante - tramite segnalazione dell'autovelox nello stesso tratto stradale di competenza, nello stesso ente, in un periodo di tempo di un'ora, è disposto il pagamento di una sola sanzione, quella più grave aumentata di un terzo se più favorevole. Siamo intervenuti anche su un altro tema importante, quello dell'abbandono degli animali. Nei primi sei mesi dello scorso anno, 242 persone sono state denunciate per aver abbandonato il proprio animale domestico. Questo provvedimento prevede l'arresto fino a tre anni se l'abbandono avviene su strada o relativa pertinenza; l'ammenda è aumentata di un terzo se il reato è commesso mediante uso di un veicolo, e la patente di guida è sospesa da sei mesi ad un anno. Basta abbandonare gli animali domestici, perché è una gravissima ingiustizia nei confronti degli animali che vivono nelle nelle case dei nostri cittadini. *(Applausi)*. Per quanto riguarda le moto, si prevede l'inserimento degli utenti delle due ruote a motore nella categoria degli utenti vulnerabili della strada. In base a questa misura, i proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie potranno essere destinati a iniziative di valore sociale e culturale volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla mobilità motociclistica. Inoltre è stata data la possibilità ai motoveicoli di cilindrata di 120 cc di circolare in autostrada e sulle tangenziali, sempre naturalmente che il conducente sia maggiorenne, ed è stato introdotto l'obbligo di installazione della terza fascia di *guardrail*, ove prevista. Grande attenzione anche alle persone con disabilità. Abbiamo voluto inserire nel codice la possibilità di aggiungere ai semafori segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e viene riservata attenzione particolare alla pavimentazione, mentre oggi assistiamo a delle realtà di assoluto degrado. Per quanto riguarda i monopattini, altro tema delicato e di attualità, il numero di incidenti, anche mortali, è purtroppo esploso. Bisognava intervenire e lo abbiamo fatto con decisione: per chi fa uso di questi mezzi abbiamo inserito l'estensione dell'obbligo del casco a tutti i conducenti, indipendentemente dall'età. Viene disposto il divieto assoluto di circolare in contromano, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile. È limitato l'ambito di circolazione dei monopattini esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore ai 50 chilometri all'ora. È disposto infine l'obbligo di contrassegno e di assicurazione del mezzo. Visto il numero di incidenti, molte volte anche con feriti gravi, prevedere l'obbligo di assicurazione e quello di avere un dispositivo di riconoscimento è assolutamente importante, dignitoso e fondamentale. Repressione, ma anche tantissima prevenzione: l'educazione stradale, che già rientra nei programmi dell'educazione civica, che abbiamo reintrodotto grazie a una legge della Lega della scorsa legislatura, sarà oggetto di corsi extracurriculari destinati agli studenti delle scuole superiori. Per tutto questo rinvolgo un doveroso e sentito ringraziamento al nostro ministro Matteo Salvini per l'impegno che sta dimostrando ogni giorno sul fronte della sicurezza delle nostre strade. Il Ministro ha consegnato al dibattito parlamentare - dobbiamo essere chiari su questo - un disegno di legge di revisione, finalmente organica, chiara e di buonsenso, del codice della strada, che non percorre la via degli interventi *spot* ideologici all'interno di decreti legge, che non hanno fatto altro che creare il caos nelle nostre strade, come purtroppo è accaduto nella passata legislatura. Dunque, dopo decenni di attesa, grazie alla determinazione del Ministro e del Governo, si è avuta la forza di aggiornare il codice della strada. Più sicurezza per gli utenti: tema tornato finalmente centrale nell'azione di questo Governo, con una riforma organica e pene più severe per i trasgressori. Lo avevamo promesso e siamo riusciti a portarlo in Aula il più velocemente possibile. Ringrazio il relatore e ringrazio anche la Commissione competente. È un messaggio di fiducia che abbiamo il dovere noi stessi di trasmettere, soprattutto ai più giovani, per onorare i tanti che purtroppo hanno perso la vita in un incidente stradale. La nostra speranza è che con questa iniziativa abbiamo anche noi mantenuto un'altra promessa fatta a tutti gli italiani: quella di garantire maggiore sicurezza sulle strade del nostro Paese. *(Applausi)*.

È un tema che tocca da vicino ciascuno di noi, che richiede una riflessione profonda e soprattutto un impegno convinto, concreto e immediato. I numeri relativi agli incidenti stradali in Italia ci danno un quadro tragico: nel solo 2022 abbiamo registrato 3.159 morti e oltre 220.000 feriti. Questo significa, per capirci, 9 morti e circa 600 feriti ogni giorno. Pensiamo alle conseguenze per le famiglie, per le comunità e per il Servizio sanitario nazionale, costretto a gestire una vera e propria emergenza nazionale. È inaccettabile che l'Italia, uno dei Paesi europei con il peggiore tasso di mortalità stradale e la minore riduzione degli incidenti mortali, non intervenga su questo. Ancora più inquietante è che ci siano tantissimi giovani tra le vittime: gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovanissimi; il 70 per cento dei sinistri avviene in ambito urbano, dove dovremmo tutti sentirci più sicuri. Dietro questi numeri ci sono vite spezzate, famiglie distrutte, sogni e speranze infranti per sempre. Allora non possiamo più parlare di incidenti come se fossero eventi casuali o inevitabili. La realtà è che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scontri causati da azioni non corrette, velocità eccessiva, distrazione, mancato rispetto delle regole. Questi sono comportamenti che possiamo e dobbiamo contrastare e l'attuale revisione del codice della strada voluta dal Governo rappresenta una gigantesca occasione persa, l'ennesima. Anzi, consiglio ai colleghi della Lega di ricordare questo al ministro Salvini, piuttosto che altro. Avevamo sperato che fosse l'inizio di un cambiamento radicale per mettere al centro la sicurezza delle persone nella nuova visione della mobilità. Purtroppo ci troviamo di fronte a un provvedimento che non affronta i problemi reali e che rischia di aggravare semmai la situazione. Questo codice limita l'autonomia dei Comuni, ostacolando interventi cruciali come le zone a traffico limitato. Noi lo avevamo fatto in Commissione con il senatore Basso, cercando di emendare il testo, lo faremo in Assemblea domani, discutendo di emendamenti che parlano di piste ciclabili, di Città 30, con una limitazione cioè della velocità a 30 chilometri orari. In molte città europee questi accorgimenti sono stati utili a salvare delle vite umane. Penso a città come la nostra Bologna, ma anche a Amsterdam, Copenaghen e Barcellona, che hanno trasformato le loro strade in spazi pubblici invece che spazi di vita e di morte. Governo invece ha scelto di seguire un modello obsoleto che rafforza la dittatura dell'automobile; non si investe infatti nella mobilità sostenibile, non si adottano misure per proteggere i pedoni e i ciclisti, non si affronta il problema della velocità e della disattenzione alla guida. Addirittura le nuove definizioni tecniche rendono più difficili interventi, come la realizzazione di piste ciclabili sicure. Noi, come Partito Democratico, abbiamo portato avanti con forza, costanza e decisione la battaglia per la sospensione della patente in caso di utilizzo dello *smartphone* alla guida, che troviamo come norma in questo provvedimento. È il primo piccolo passo. Ogni giorno, infatti, decine di persone muoiono o rimangono ferite perché qualcuno guarda uno schermo anziché la strada. Stare sei o sette secondi con lo sguardo su un telefono, anche a 50 chilometri orari, significa fare 100 metri a occhi chiusi; a velocità più alta, tutto questo diventa pura follia. Chi uccide qualcuno perché era in diretta *social* o scriveva un messaggio, non è una persona sbadata, ma si macchia di un atto senza rimedi. Eppure, per casi del genere, il Governo non ha voluto introdurre un'aggravante per l'omicidio stradale, nonostante le promesse del ministro Salvini, una delle tante di propaganda che ha fatto prima di portare questo provvedimento alla luce e alla discussione in Parlamento. *(Applausi)*. Ciò è inaccettabile soprattutto per il futuro delle nuove generazioni. Questa revisione del codice della strada costituisce un pesante arretramento perché ci mette davanti a maggiore velocità, a minori controlli, a tutele ridotte al lumicino rispetto ai pericoli e di fronte alle esigenze dei più fragili. Inoltre, il testo determina più tolleranza per chi ignora divieti, più punizione per chi sceglie mezzi meno inquinanti e meno autonomia per i sindaci. Insomma il centrodestra conferma, a discapito dei cittadini, la sua predilezione per fare liberi tutti, la sua avversione per chi governa i territori, la sua ostilità per la mobilità sostenibile e la volontà di imporre modelli di vita che generano consenso, disparità e danni collettivi. Il costo sociale degli incidenti stradali in Italia ammonta a 18 milioni di euro l'anno; una cifra enorme che potrebbe essere investita in infrastrutture, tecnologie e campagne di sensibilizzazione per salvare le vite umane. Purtroppo il dibattito pubblico, invece, si concentra su questioni marginali, come la classifica dei Comuni che fanno più multe, senza affrontare il problema alla radice. Dobbiamo semmai iniziare a pensare a come utilizzare le nuove tecnologie a nostra disposizione per migliorare la sicurezza. Penso alle notifiche digitali e immediate delle multe che aiuterebbero anche i cittadini a collegare il comportamento scorretto alla sanzione, favorendo anche un cambiamento culturale da parte dei cittadini. Penso a dispositivi obbligatori per eliminare gli angoli ciechi nei mezzi pesanti; una misura che il Governo ha inspiegabilmente bocciato e su cui avevamo presentato delle proposte. Penso ai simulatori di guida e alla formazione permanente, che potrebbero fare la differenza. La sicurezza strada stradale non può essere separata dalla mobilità sostenibile; investire nella ciclabilità, nel trasporto pubblico locale, nella riduzione del traffico privato non è solo una questione ambientale, ma è una questione di sicurezza e di qualità della vita. Questo Governo ha scelto però di andare nella direzione opposta, riducendo le tutele per i pedoni e i ciclisti, ostacolando la progettualità delle amministrazioni locali. Le nostre città devono diventare spazi dove tutti, indipendentemente dall'età o delle condizioni fisiche, possono muoversi in sicurezza. Dobbiamo ripensare lo spazio pubblico, ridurre la velocità nei centri urbani e incentivare modalità di trasporto più sicure e meno inquinanti. Questo è il futuro della mobilità. È una battaglia che il Partito Democratico continuerà a portare avanti, specie di fronte a una miopia cronica del Governo. Alcuni interventi che oggi abbiamo ascoltato in discussione generale, dimostrano di essere totalmente al di fuori della realtà, necessari solo per difendere un testo della propria parte politica. *(Applausi)*. La sicurezza stradale non è un tema di destra o di sinistra, ma è una questione di responsabilità collettiva. Come legislatori, abbiamo il dovere di mettere al primo posto la vita e la sicurezza delle persone, ma questo significa fare scelte coraggiose, investire nelle tecnologie e nelle infrastrutture, così come lavorare per una mobilità più sostenibile e inclusiva. Serve, però, l'impegno di tutti, perché la sicurezza stradale è una battaglia che riguarda ciascuno di noi e non possiamo permetterci di aspettare ancora. Ogni giorno perso significa altre vite spezzate, altri sogni infranti; abbiamo il dovere morale e politico di fermare questa strage silenziosa.

entro domani approveremo la prima vera riforma del codice della strada in trentadue anni. Rimarco: trentadue anni. Dopo tutto questo tempo, c'era la necessità di intervenire in maniera sistematica, aggiornando il corpo normativo alle esigenze e alle problematiche non ancora risolte della sicurezza stradale. Avrei voluto invitare tutti ad evitare sterili polemiche, ma sono evidentemente in ritardo. Tuttavia, permettetemi di dire che, se è vero che un provvedimento è sempre migliorabile, è anche vero che non si può rinviare continuamente in attesa dell'atto perfetto. È a causa di tale ragionamento se gli italiani hanno aspettato decenni, ad esempio, per la riforma fiscale. Questo provvedimento, dunque, è un'ulteriore dimostrazione che questo Governo e questa maggioranza vogliono essere ricordati per le cose fatte e non per le parole spese. Sulla sicurezza stradale, molto è stato fatto e molto c'è da fare, ne siamo consapevoli. Penso di non poter essere smentito se affermo che questo disegno di legge è il frutto di un intenso lavoro prima alla Camera e poi anche qui in Senato, che ha interessato mesi di attività parlamentare, lavoro in cui si è dato spazio a tutte le parti sociali e a tutti i Gruppi parlamentari. Molti emendamenti meritevoli di attenzione sono stati trasformati in ordini del giorno e costituiranno la base per approfondimenti in sede di attuazione della delega. Vorrei ricordare alcuni di questi ordini del giorno, sia della maggioranza, sia dell'opposizione, i quali impegnano il Governo ad introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori e lavoratori critici, come ad esempio il trasporto su strada, o ad introdurre deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, ad esempio per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato, quali i mezzi agricoli. Anche in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi sono stati accolti ordini del giorno che portano all'attenzione del Governo la problematica della sicurezza sulle strade extraurbane (mi riferisco Questo significa che il nuovo codice della strada non sarà perfetto, ma è perfettibile. Il Governo non si tira indietro nel dare al Paese la legislazione migliore con il contributo di tutti. Ne è esempio il decreto legislativo presentato proprio nei giorni scorsi sulle disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti, arricchito, dunque, tenendo conto delle osservazioni arrivate a seguito del confronto con le categorie. La dialettica, però, non può e non deve essere una scusa per non decidere mai. Gli italiani hanno il diritto di avere un nuovo codice della strada oggi e non domani, un codice che sia aggiornato e che vada incontro alle necessità di sicurezza stradale che i cittadini ci chiedono, necessità necessità che sono mutate in oltre trent'anni. Le norme, quindi, devono essere adattate ai tempi. È un provvedimento che guarda sia alla prevenzione, con nuove norme sull'educazione stradale, sia alla dissuasione dal porre in essere comportamenti pericolosi, attraverso l'inasprimento delle sanzioni. Tutti sappiamo, infatti, ma forse è bene ripeterlo, che in Italia come nel resto d'Europa, gli incidenti stradali non sono diminuiti. L'età media dei cittadini coinvolti si è abbassata e sappiamo tutti - ma è bene ricordare - anche questo, ovvero che le principali cause degli incidenti stradali sono l'alcol, le sostanze stupefacenti, la distrazione e la velocità. Quando analizziamo questo provvedimento con obiettività, ci rendiamo conto che incide proprio su questi fattori, che sono le principali cause d'incidente, secondo l'approccio del sistema sicuro, che mira a riformare la politica in materia di sicurezza stradale, concentrandosi sulla prevenzione. Le modifiche sono improntate al principio, invocato da tempo dall'Unione europea, della tolleranza zero nei confronti di tutti i conducenti che guidano avendo abusato di alcol o che si mettono alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti:

È per questo che all'articolo 1 si inaspriscono le sanzioni e le pene verso chi guida in stato di ubriachezza e si sopprime il riferimento allo stato di alterazione psicofisica in relazione all'assunzione di stupefacenti. Questo consentirà di sanzionare la guida anche dopo aver assunto droghe, superando la difficoltà di dimostrare il nesso tra assunzione della sostanza e l'effetto dell'alterazione psicofisica. merita anche una menzione l'introduzione della sanzione della sospensione breve della patente di guida. L'articolo 3 prevede una sanzione aggiuntiva rispetto alla decurtazione dei punti quando vengono commesse alcune infrazioni, tassativamente elencate. Si tratta anche in questo caso di norme di deterrenza per infrazioni che potrebbero sembrare minori, ma che comunque mettono in pericolo la sicurezza stradale, quali il mancato rispetto del segnale di senso vietato e di divieto di sorpasso, la circolazione contromano, la mancata precedenza, il mancato rispetto della segnalazione del semaforo o dell'agente del traffico che vietino la marcia; è anche prevista la sospensione breve per chi guida guardando il cellulare. Non possiamo, infatti, nasconderci che la distrazione al volante è una delle maggiori cause di incidenti stradali. Il testo è ricco di novità che sarebbe lungo esaminare, ma che hanno lo scopo di assicurare una maggiore sicurezza stradale, introducendo la previsione di ulteriori obblighi relativi all'esercitazione alla guida per coloro che vogliono prendere la patente (articolo 7).

In dettaglio, la disposizione prevede che, nel caso di violazioni reiterate del limite di velocità entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario, non vi sia il cumulo materiale delle sanzioni, ma il cumulo giuridico, così come previsto dall'articolo 198 del codice della strada. Molti, anche questa sera, hanno invocato lo scandalo su questa disposizione perché si agevolerebbero le infrazioni; in realtà, invece, la norma fissa parametri certi per quello che oramai è un indirizzo della giurisprudenza. Infatti, già da molto tempo le corti italiane considerano unica la condotta di chi supera velocità rilevate da più autovelox su un unico tratto di strada per un certo periodo di tempo. Il nuovo articolo 142 del codice della strada oggi stabilisce quando il tratto di strada può considerarsi unico, ovvero quando appartiene allo stesso ente, e quanto tempo dopo l'infrazione la condotta non si può considerare unica, ovvero un'ora dall'infrazione. Altre norme meriterebbero attenzione, come ad esempio l'articolo 13, che adegua le somme a compenso per le operazioni di revisione dei mezzi pesanti e di esame di patente che vengono espletate dai dipendenti in conto privato o in orario straordinario. Pensate, colleghi, che la norma non era mai stata modificata dal 1986. Non dobbiamo dimenticare - e questo provvedimento

all'articolo 14, prevede nuove norme per garantire la sicurezza di coloro che usano questi mezzi di trasporto, ad esempio per chi si muove in monopattino, con l'obbligo dell'uso del casco, l'apposizione di una targa identificativa, l'installazione di una freccia direzionale, la stipula di un'assicurazione. C'è chi vede le nuove norme come un ostacolo alla diffusione della mini mobilità, ma non è così: sono norme a tutela della sicurezza di chi utilizza questi mezzi. È una norma giusta pretendere che le piste ciclabili siano ben separate e non solo da una striscia a terra, che evidentemente non è adatta a salvaguardare la sicurezza di chi utilizza biciclette, soprattutto quando la sede stradale non è abbastanza ampia. Non possiamo negare, perché è accaduto in tutte le città, piccole o grandi che siano, dal Nord o al Sud, che siano proliferate corsie preferenziali per i ciclisti, ovvero semplici delimitazioni di una parte della carreggiata, spesso su strade che non sono sufficientemente ampie, spacciate per piste ciclabili. Tutto questo solo per dire che si è contribuito alla mobilità sostenibile. Invece, molto spesso queste corsie preferenziali sono trappole per i ciclisti. Quando parliamo di tutela della sicurezza, non possiamo barattarla con false ideologie. I ciclisti sono utenti della strada, ma sono utenti vulnerabili e nei loro confronti vanno utilizzate maggiori cautele. È proprio per questo che è una norma di civiltà

dà una stretta a tutti quei comportamenti che possono generare incidenti stradali. Ci viene contestato, da quando questa maggioranza è stata eletta e da quando il Governo si è insediato, di avere esautorato il Parlamento della sua funzione legislativa. Io ritengo, invece, che non sia mai stato così e l'*iter* del nuovo codice della strada ne è l'esempio lampante. Certamente potranno esserci integrazioni, ma evidentemente una materia così importante e complessa necessita di una trattazione organica da parte del Governo, che posso garantire non si sottrarrà al confronto durante l'attuazione della delega che gli stiamo conferendo. Torno a ribadirlo: non si può e non si deve rimanere sempre nel limbo delle proposte, del "ci vorrebbe questo o quest'altro", né si possono perdere anni nella discussione. L'Italia ha bisogno di riforme. Sono decenni che nessun Governo prende su di sé la responsabilità di adeguare le normative ai nuovi contesti e alle nuove esigenze degli italiani. Questo Governo lo fa. Del resto, questo è il primo Governo politico che l'Italia ha in decenni. Del resto, questo è il Governo dei fatti.

Signora Presidente, questo intervento è per porre l'attenzione rispetto ad una grave crisi occupazionale che in questi giorni sta maturando il suo epilogo, che noi speriamo sin d'ora sia positivo. Stiamo parlando della crisi occupazionale della Beko Europe, la quale ha visto un tavolo di confronto il 7 novembre, quando l'azienda ha rappresentato la volontà di una revisione delle attività produttive, produttive, che vanno a coinvolgere alcuni stabilimenti in Italia ove vi sono migliaia di lavoratrici e lavoratori interessati. Nello specifico, stiamo parlando dei siti produttivi di Cassinetta, nella provincia di Varese, di Siena, di Comunanza e di altri. Ebbene, noi oggi vogliamo esprimere vicinanza allo stato d'animo di tutte quelle donne, tutti quegli uomini, tutte quelle famiglie, che vivono questa ennesima incertezza. Ennesima perché, solo lo scorso 2 aprile, la Whirlpool ha ceduto a Beko una serie di stabilimenti, una serie di unità produttive e di settori produttivi e, a distanza di pochi mesi, oggi ci troviamo all'ennesima crisi, negli stessi stabilimenti, nelle stesse unità produttive, dove si parla di dismissione. Noi ci domandiamo oggi anche quali siano state le garanzie nei tavoli di confronto che si sono svolti ad aprile, con le quali il Governo ha acconsentito a questo trasferimento di proprietà, e perché non abbia esercitato fino in fondo i poteri speciali, la cosiddetta *golden power*, per garantire che vi fosse una continuità aziendale e che non fosse solamente un ipotetico passaggio di mano, che poi oggi ci porta nelle medesime condizioni di partenza. Noi facciamo questo intervento perché domani si tiene al Mimit, alla presenza del ministro Urso, l'ennesimo tavolo di confronto. Noi auspichiamo che non sia l'ultimo tavolo di confronto, ma che domani emerga per quelle lavoratrici e quei lavoratori una prospettiva di lavoro e di dignità per loro stessi e per le loro famiglie. Questo anche per il sistema produttivo italiano e per la manifattura che, pezzo dopo pezzo, il nostro Paese vede

i recenti omicidi di Emanuele Tufano, Santo Romano e Arcangelo Correra, che hanno profondamente scosso la città di Napoli, non sono solo episodi di cronaca nera, ma volti che ci guardano, storie spezzate che ci chiedono giustizia. È un allarme che risuona, più che nelle strade di Napoli, nelle coscienze di tutti noi italiani. Mi chiedo, anzi ci chiediamo, perché siamo arrivati a questo punto, perché i nostri giovani si sentono così persi e così privi di punti di riferimento. Ammettiamolo, la risposta è chiara: viviamo in una società in cui lo Stato, spesso assente, lascia che le città, al calar delle tenebre, diventino terra di nessuno. In questo vuoto i nostri ragazzi cercano risposte, ma trovano soltanto il richiamo seducente della violenza e della criminalità. Che cosa possiamo fare per restituire loro la speranza? Come possiamo garantire che la loro voce non venga soffocata dal rumore della paura e dall'angoscia di non vedere il futuro? È nostro dovere restituire loro la possibilità di sognare e guardare al loro futuro con fiducia. È però fondamentale che lo Stato non intervenga solo con risposte di emergenza e misure repressive. Ormai è giunta l'ora di orientarli nel medio e lungo termine, investendo nell'istruzione affinché, attraverso la cultura e con la formazione, si creino gli anticorpi per realizzarsi come individui. Occorre creare un ambiente in cui i nostri ragazzi possano sentirsi parte di una comunità che li accoglie, li indirizza e li sostiene. Onorevoli colleghi, non c'è altra strada se non un cambiamento radicale, che si può ottenere introducendo l'educazione emotiva nelle scuole, cioè dare un'ora di lezione in più. A tal fine, sto lavorando a un disegno di legge con l'obiettivo di implementare l'educazione emotiva nelle scuole italiane, incrementando il monte ore scolastiche e istituendo un fondo preposto preposto ad aggiornare gli insegnanti almeno ogni due anni, affinché siano in grado di insegnare competenze emotive e sociali ai loro studenti. L'intento è di formare non solo studenti, ma cittadini consapevoli, capaci di affrontare le sfide della vita con empatia, rispetto di genere e responsabilità individuali. Onorevoli colleghi, la criminalità non è solo un nemico esterno, è un nemico che cresce dentro le nostre comunità, alimentato dalla mancanza di opportunità di lavoro, dalla disillusione in un miglioramento di vite che si realizza con la rinuncia e l'abbandono della scuola. Per questo, ogni giorno che passa senza un intervento deciso dello Stato è un giorno in cui altri ragazzi rischiano di perdersi e di essere strappati alla vita. Pertanto, è tempo di agire e costruire un sistema educativo inclusivo che accolga ogni giovane, mettendosi in ascolto per cogliere le istanze dei ragazzi e delle loro famiglie. Dobbiamo rendere le nostre scuole luoghi dove i valori della legalità, della solidarietà e della giustizia possano riaffermarsi. Dobbiamo lavorare insieme, come comunità e istituzione, per costruire un futuro in cui ogni giovane possa sognare, crescere e investire in territori in cui la vita e la speranza possano prevalere sulla violenza e sulla disperazione. Onorevoli colleghi, abbiamo il dovere di non lasciare che la storia di Emanuele, Santo e Arcangelo sia solo un triste capitolo di cronaca. Anzi, facciamo in modo che il loro sacrificio diventi un faro che ci spinge a lottare per un futuro in cui le pistole siano sostituite da libri, i coltelli dalla cultura e i comportamenti violenti da un profondo rispetto per tutti gli esseri umani.

una sanguinosa dittatura sprezzante di qualsiasi diritto, di qualsiasi libertà, di qualsiasi democrazia; e l'Ucraina per quello che è, la coraggiosa frontiera di quei diritti, di quelle libertà, di quella democrazia che chiamiamo Europa. Ora più che mai, signor Presidente, gli ucraini hanno urgenza del nostro sostegno e aiuto, militare innanzitutto, politico, economico. Penso a cosa significherà la ricostruzione, anche in termini di fondi da stanziare, perché la Russia venga costretta a pagare per l'incalcolabile devastazione che ha causato. Ora più che mai dobbiamo sapere che quello che non solo è accaduto, ma che accade ogni giorno nelle loro città ancora oggi (bombardamenti, distruzione, morti di civili, sangue), è il prezzo che un intero popolo sta pagando non solo per la sua, ma per la nostra libertà; non solo per la sua, ma per la nostra democrazia; non solo per i suoi valori, ma per i nostri valori di italiani e di europei. Ora più che mai, signor Presidente, *Slava Ukraïni*.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

Grazie